Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze*: «Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 maggio. Al primo punto dell'ordine del giorno di oggi è stata inserita l'informativa del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla febbre suina. Successivamente potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi per 5 minuti ciascuno. Si passerà poi alla discussione del disegno di legge collegato sul federalismo fiscale, che proseguirà nelle due sedute convocate per la giornata di domani. Le dichiarazioni di voto, con trasmissione diretta televisiva, avranno luogo domani alle ore 19. Seguirà il voto finale con la presenza del numero legale. La discussione del disegno di legge collegato in materia di internazionalizzazione imprese ed energia, già prevista già prevista dal precedente calendario per la settimana corrente, avrà inizio nella seduta pomeridiana di martedì 5 maggio. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi. Nel corso della prossima settimana sarà inoltre discussa la mozione Sbarbati e altri sulla promozione della cultura. Nella seduta pomeridiana di giovedì 7 maggio si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla febbre suina». Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti.

è endemico nella popolazione suina mondiale e rappresenta in tale specie una causa frequente e primaria di patologia respiratoria. Attualmente sono endemici nella popolazione suina in Europa i tre sottotipi virali H1N1, H3N2 e H1N2. Il 24 aprile 2009 giungevano sia dagli Stati Uniti che dal Messico conferme di casi di infezione umana da virus influenzale suino H1N1. Ha ragione, tuttavia, la commissaria europea alla salute Androulla Vassiliou nel definire questa patologia "nuova influenza", in quanto, come la stessa commissaria ha spiegato, la definizione sinora usata «poteva indurre in errore, dato che la carne suina, se cotta, non presenta alcun rischio per la salute. Il nuovo nome» - dice ancora la commissaria - «è stato scelto per non produrre un effetto negativo sull'industria del settore». Per quanto riguarda lo stato di diffusione della malattia a livello mondiale, inizialmente, sono stati notificati dagli Stati Uniti sette casi, riscontrati negli Stati del Texas e della California, alcuni dei quali riguardavano soggetti che si erano recati precedentemente in Messico. Nello stesso 24 aprile il Governo del Messico ha riportato informazioni in ordine a focolai di infezioni umane di virus influenzali A/H1N1 riguardanti almeno 3 aree: Distretto federale del Messico, San Luis Potosi (Messico centrale) e Mexicali in prossimità dei confini con gli Stati Uniti. Su campioni biologici dei casi messicani inviati al laboratorio di virologia di Winnipeg (Canada) è stata confermata l'infezione da virus influenzale suino A/H1N1, con individuazione, in alcuni di questi, di una sequenza genetica identica a quella dei virus suini A/H1N1 A/H1N1 isolati dai casi americani. La maggior parte dei casi è stata osservata in giovani adulti precedentemente in buona salute. Si tratta di un dato inusuale, in quanto l'influenza solitamente colpisce con maggiore frequenza le persone molto anziane e i bambini. Gli eventi segnalati hanno destato notevole preoccupazione, in considerazione dei casi di infezione umana con un virusinfluenzale animale, della diffusione geografica di più focolai epidemici dovuti allo stesso ceppo virale in diverse comunità e dell'insolita fascia di età coinvolta.

in Messico la maggiore sorveglianza ha portato ad evidenziare, dal 17 al 26 aprile, 1.455 casi di sindrome similinfluenzale (ILI), con oltre 90 decessi. Questi casi sono stati registrati in 24 dei 32 Stati del Messico, ma per la maggior parte risultano essere concentrati nel Distretto federale (in cui si trova la capitale nello Stato di Mexico e in San Luis Potosi. Per maggiore precisione, va detto che i casi accertati da nuovo virus dell'influenza di tipo A/H1N1, confermati in laboratorio, sono 26 ed i decessi sicuramente attribuiti a tale infezione sono 7.

(fase in cui un virus influenzale riassortante animale o umano-animale causa casi sporadici o piccoli focolai di malattia tra l'uomo, ma non si è ancora verificata una trasmissione da uomo a uomo sufficiente per sostenere focolai epidemici a livello di comunità) alla attuale fase 4 (caratterizzata da una trasmissione accertata da uomo a uomo di un virusinfluenzale riassortante animale o umano-animale in grado di causare focolai a livello di comunità). La capacità di provocare epidemie estese in una comunità, infatti, segna un significativo passaggio nel rischio di pandemia. Alla data del 27 aprile la sorveglianza accresciuta raccomandata dall'OMS ha portato ad ha portato ad identificare casi di influenza umana da virus A/H1N1 anche in altri Paesi: in particolare 6 casi confermati sono stati segnalati dal Canada, mentre i casi confermati negli USA sono 40. Sia i casi confermati in Canada sia quelli degli USA hanno presentato sintomi influenzali modesti e non si è riscontrato tra loro alcun decesso. La situazione è diversa in Messico, con numerosi decessi, ancora sotto indagine per una definitiva conferma di laboratorio sulla loro natura. Come detto, tra questi, i casi confermati, nel periodo compreso tra il 17 e il 24 aprile, sono stati 26, tra cui 7 casi mortali. Al momento in Italia sono stati segnalati alcuni casi (esattamente 11 alle ore l6 di oggi) considerati sospetti sulla base del criterio epidemiologico (recente soggiorno in aree affette), ma le indagini di laboratorio hanno escluso che si trattasse di casi di influenza da ceppo suino A/H1N1. Per quanto riguarda la strategia di contrasto intrapresa dal Ministero, sottolineo preliminarmente che il Paese è in grado di fronteggiare sicuramente il trattamento dei casi che dovessero inizialmente verificarsi sul territorio nazionale nazionale e che il Ministero, pur non sussistendo le condizioni idonee a destare un diffuso stato di allarme nei cittadini, non sottovaluta comunque la rilevanza sanitaria del fenomeno. Il Ministero ha adottato tutte le iniziative necessarie a fronteggiare eventuali emergenze. In tale prospettiva ha innanzitutto attivato un'unità di crisi *ad hoc*, presieduta dal sottosegretario professor Ferruccio Fazio, e composta da rappresentanti del Ministero, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco e del mondo scientifico. La strategia complessiva si basa sull'interazione sinergica di tre reti: quella deputata alla sorveglianza epidemiologica delle sindromi similinfluenzali ovvero la rete INFLUNET, che si avvale di circa 1.000 medici sentinella sparsi su tutto il territorio; quella deputata alla sorveglianza virologica, che si avvale di 25 laboratori accreditati dal laboratorio di riferimento nazionale presso l'Istituto superiore di sanità; infine, la rete di degenze protette, costituita dai reparti di malattie infettive dotati di stanze di isolamento. Sul piano dell'informazione, al fine di fornire adeguate risposte alle continue domande dei cittadini sugli eventuali rischi connessi alla diffusione della «nuova influenza», è stato attivato un servizio di informazione telefonica alla popolazione generale ed in particolare ai viaggiatori. Già da oggi sono attive, dalle ore 8 alle ore 20, 8 linee di risposta diretta al cittadino, con il numero verde 1500. Per quanto riguarda, inoltre, le misure di prevenzione adottate dalla Direzione competente del Ministero, si è provveduto ad attivare gli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (i cosiddetti USMAF) ai fini di profilassi internazionale. È stato in particolare predisposto un modello di *poster* informativo sulla "nuova influenza", sul facsimile di quelli a suo tempo usati per l'influenza aviaria, da esporre nei contesti portuali ed aeroportuali per una più capillare informazione del pubblico. Sono state già adottate le necessarie iniziative per la distribuzione dei foglietti informativi per i viaggiatori, avvalendosi della collaborazione dell'ENAC, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e delle compagnie aeree e di navigazione. Le misure richieste per aeromobili e navi sono le seguenti. Per gli aeromobili: trasmissione obbligatoria all'Ufficio sanitario dell'aeroporto (cioè all'USMAF) all'USMAF) della parte sanitaria della dichiarazione generale di aeromobile, debitamente compilata per ciò che concerne le condizioni di salute di passeggeri e componenti di equipaggio. Per le navi: esclusione del rilascio della libera pratica via radio a qualunque nave abbia toccato porti delle aree affette. La richiesta scritta di libera pratica sanitaria dal comando di bordo deve essere trasmessa Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 232. È stata avviata una più capillare ricognizione dei voli e delle linee marittime passeggeri in arrivo dal Messico, dagli Stati Uniti e dal Canada, nonché la distribuzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) per le esigenze di tutela sanitaria del personale USMAF. Gli USMAF, da parte loro, hanno inviato comunicazioni ai soggetti e alle amministrazioni operanti in ambito portuale e aeroportuale e stanno verificando presso le autorità sanitarie locali la disponibilità di posti letto in reparti di malattie infettive. Al fine di condividere con le Regioni le misure da adottare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale per fronteggiare tale emergenza, si svolgerà domani un incontro con i rappresentanti delle stesse. A livello internazionale sono state attivate diverse iniziative, fra le quali la convocazione, da parte del direttore generale dell'OMS, del comitato di emergenza per il regolamento sanitario internazionale dello stesso organismo. Inoltre, anche a livello di Unione europea sono state adottate diverse iniziative, tra cui audio-videoconferenze giornaliere alle quali partecipano gli Stati membri,

dell'Unione europea. L'Italia, nella funzione di Paese incaricato della Presidenza G8, ha avviato una consultazione con gli otto Paesi industrializzati ed i cinque emergenti per rafforzare il coordinamento internazionale. I vaccini di cui l'Italia attualmente dispone sono purtroppo inefficaci per fronteggiare l'influenza da nuovi virus di tipo A H1N1, ma tale virus si è peraltro mostrato sensibile agli antivirali oseltamivir e zanamivir. A proposito di vaccini, ovviamente nel mondo non esistono in questo momento vaccini efficaci. Le scorte invece degli antivirali che ho citato, ai quali il virus risulta sensibile, sono stoccate presso questo Ministero e ammontano a circa 40 milioni di dosi, di cui circa 30 milioni di dosi di farmaco oseltamivir (Tamiflu) e circa 10 milioni di dosi di farmaco zanamivir (Relenza). Per prolungare la durata dell'efficacia del principio attivo oseltamivir, questo è stato acquistato soprattutto in forma di polvere, la cui durata è di 10 anni (mentre quella del prodotto incapsulato (mentre quella del prodotto incapsulato è di 5 anni). Una scorta di 60.000 dosi di Tamiflu, pronte per l'uso, è comunque già disponibile e va ad aggiungersi al farmaco Relenza (un milione di dosi) già pronto per l'uso. Per il trattamento dei casi di influenza occorre un ciclo di 10 dosi del farmaco a persona (2 capsule per 5 giorni). Ad ogni modo, ben prima dell'inizio della crisi generata dall'epidemia in atto, questo Governo pianificato il piano per l'incapsulamento dell'oseltamivir in polvere a seguito di un accordo stipulato nel dicembre 2008 con l'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze. Ricordo, in ogni caso, che questa polvere peraltro può essere assunta, in estrema emergenza, in soluzione liquida. Per quanto riguarda la congruità delle scorte antivirali, occorre sottolineare che la valutazione del fabbisogno di farmaci antivirali si basa su una serie di assunzioni e considerazioni fondate su scenari possibili da diffusione di infezioni da virus dell'influenza aviaria A/H5N1. Questi indicatori sono: la proporzione di popolazione che si potrebbe ammalare; il fatto che gli antivirali attualmente disponibili appartengono alla classe degli inibitori della neuraminidasi che non curano completamente l'influenza ma ne abbreviano il decorso clinico e quindi riducono la contagiosità del singolo caso; il fatto, ancora, che tali antivirali sono efficaci solo se assunti entro 48-72 ore dall'inizio dell'infezione e quindi richiedono una tempestiva somministrazione. L'utilizzo di tali antivirali viene previsto a scopo preventivo, somministrando l'antivirale ai contatti sicuramente esposti ad un caso contagioso confermato di influenza pandemica (questo uso è particolarmente importante nelle fasi iniziali della pandemia in cui tutti gli sforzi sono concentrati nel controllo della diffusione), diffusione), ed a scopo terapeutico per ridurre e mitigare la durata della sintomatologia nei casi in cui si temono complicazioni importanti. Si deve, peraltro, ricordare che i modelli sviluppati dall'Istituto superiore di sanità hanno evidenziato anche il contributo di altre misure di prevenzione oltre agli antivirali. Basandosi sulle assunzioni descritte, la quantità di antivirale disponibile appare dunque sufficiente per affrontare l'eventuale manifestazione di casi di pandemia in Italia. Ulteriore riduzione del numero dei casi è ottenibile mediante l'adozione contemporanea di altre misure di prevenzione nella comunità come il distanziamento sociale e, successivamente, la vaccinazione. Pertanto, ritengo doveroso sottolineare che gli antivirali sono uno strumento che insieme alle altre misure come, ad esempio, una corretta igiene sanitaria che come è noto in Italia è più robusta che in Paesi come il Messico - può contribuire a limitare il diffondersi dell'infezione. Per completezza e al fine di meglio valutare la congruità delle scorte in Italia, ed anche per evitare stucchevoli e infondatissime polemiche che generano allarme non giustificato, ritengo utile riportare i dati di stoccaggio relativi ad altri Paesi: negli Stati Uniti 50 milioni di dosi, in Francia 30 milioni di dosi, nel Regno Unito 30 milioni di dosi, in Spagna 10 milioni di dosi e in Austria 4 milioni di dosi. situazione contingente, dell'influenza suina e del percorso per arrivare al vaccino, non sono attualmente disponibili, in nessuna parte del mondo, vaccini antinfluenzali specifici per questo nuovo virus di tipo A/H1N1. sono già in corso contatti tra il Ministero e i principali produttori, in grado di sviluppare il vaccino una volta che l'OMS avrà reso disponibile il ceppo virale responsabile della nuova infezione, per orientarsi su una strategia nazionale in merito. Ferma restando dunque la possibilità concreta di avvalersi di farmaci antivirali per la gestione di eventuali casi che possano manifestarsi in Italia, ritengo comunque utile ricordare in questa sede il percorso necessario per arrivare alla produzione di un vaccino per l'influenza suina. Il virus deve essere prima isolato e poi caratterizzato, cioè ne viene individuata la sequenza genetica; l'Organizzazione mondiale della sanità consegna il virus isolato ai produttori di vaccini; di vaccini; la stessa OMS, gli Stati e le aziende produttrici decidono la strategia produttiva e, come ho detto, noi siamo già pronti a ciò. Individuata infine la strategia produttiva occorre che il vaccino superi le prove tecniche di efficacia e tollerabilità. Vorrei infine sottolineare il merito che hanno avuto alcuni operatori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che, nel corso del 2006, hanno resa pubblica la necessità di condividere e diffondere, nell'ambito della comunità scientifica internazionale, le sequenze geniche dei virus dell'influenza aviaria. A seguito di tale iniziativa nel 2008 è nato il «*Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data*» che rappresenta un *network* mondiale finalizzato a condividere dati scientifici, in modo tale che le sequenze genetiche dei virus dell'influenza aviaria siano raccolte e disponibili in tutto il mondo per comprendere più adeguatamente le origini, i meccanismi di patogenicità e le caratteristiche in generale dei virus. Nello stesso *database* sono stati riversati dai *Centers for Desease Control* di Atlanta le sequenze geniche del virus dell'influenza suina e, pertanto, tale *network* sta svolgendo un ruolo cruciale nella ricostruzione dell'identikit genetico di tale virus. Per quanto riguarda infine gli aspetti di sanità veterinaria, a seguito dell'attività di sorveglianza effettuata dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, in Italia, al momento, non esiste alcuna evidenza di circolazione dello stipite virale messicano. I virus circolanti in Italia non presentano analogia strutturale con il virus H1N1 riscontrato in Messico. L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che il rischio di infezione correlato al consumo di carne suina e prodotti derivati è irrilevante. Infatti, la cottura della carne determina l'inattivazione virale, così come la «maturazione» cui vengono sottoposti gli insaccati. Peraltro non vi sono importazioni in Italia di suini, non solo dai Paesi sopra indicati, ma di fatto da tutti i Paesi terzi. Alla luce della situazione complessiva e delle iniziative adottate a livello nazionale e internazionale, si sottolinea quindi che la situazione sanitaria è costantemente monitorata dagli organismi di riferimento a livello centrale e territoriale. In sintesi, come ho più volte ripetuto insieme al collega sottosegretario Fazio in questi giorni, non c'è nessuna sottovalutazione, ma allo stesso tempo nessuna ragione di allarmismo ingiustificato. Signora Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, ringraziandovi per questa ampia informativa, desidero sottolineare, con un breve intervento a nome del mio Gruppo, l'efficienza dell'apparato sanitario italiano messo in moto in questa occasione,

sia dal punto di vista scientifico, quanto all'identificazione del virus, ai laboratori aperti e attivi sul territorio, alla presentazione di norme precise e alle scorte del farmaco efficace. certo che la globalizzazione non riguarda solo i sistemi finanziari, ma anche le malattie e soprattutto la prevenzione e le cure. Devono dunque essere pensate e progettate a livello mondiale iniziative comuni: una comunicazione tardiva della malattia, come quella verificatasi in Messico, può essere pericolosa non solo per quella Nazione. Signor Ministro, la possibilità che la malattia si stia diffondendo e stia arrivando in Europa esiste. esiste. Nella nostra piccola Valle d'Aosta, che presenta diverse frontiere e molte porte di entrata, viviamo una preoccupazione sanitaria particolare. Vi esortiamo dunque, signor Ministro e signor Sottosegretario, a non abbassare la guardia, ad insistere

Non si tratta di allarmismi, perché autorevoli esponenti del campo medico e scientifico sono i primi a sottolineare la necessità di tenere molto alta l'attenzione, in quanto il fenomeno non è ancora esattamente quantificabile. Ha ben ragione il professor Massimo Galli, docente di malattie infettive dell'Università di Milano, quando dice che non si può prevedere nulla: potremo trovarci in una situazione di massima gravità

forse sarebbe stata più completa ed esaustiva se avesse informato il Parlamento sulla

Così come avremmo voluto avere qualche ulteriore rassicurazione non solo sulla sufficienza della quantità delle dosi, che come giustamente ha ricordato il Ministro è ad un livello superiore ad altri Paesi,

della preparazione del farmaco, come demandato all'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze. Questo perché

basate soltanto sull'uso di volantini contenenti consigli per i viaggiatori, non debbano essere ulteriormente appoggiate e sostenute da una campagna di sensibilizzazione che, senza stimolare allarmismi, come ha sottolineato il Ministro, possa però fare una maggiore opera di informazione. Sulla base di questi elementi, riteniamo che il Ministero della salute debba tenere molto alta la guardia su questo problema, perché è bene essere estremamente prudenti rispetto ad una situazione di sanità pubblica

soprattutto ci rassicura la metodologia con cui il cordone è stato costruito, soprattutto a livello aeroportuale. Infatti, il virus non può arrivare da solo, ma deve venire attraverso qualche individuo infetto.

più assilla la cittadinanza e quanto più rischierebbe di rovinare alcuni settori della nostra economia, come in un passato recente è avvenuto per altre influenze (ultima delle quali è stata

nell'esortare ulteriormente il Ministero a non abbassare la guardia e soprattutto a continuare con questa corretta e lineare informazione,

questa informativa, che è necessaria a causa del continuo evolversi e susseguirsi di notizie ed indiscrezioni che certamente stanno destando non poche preoccupazioni tra i nostri concittadini. Abbiamo chiesto subito, come Partito Democratico, un intervento a livello istituzionale, poiché i giornali degli ultimi giorni e le notizie che man mano si susseguono parlano di un'influenza che comunque va oltre i confini del Messico ed è ormai arrivata in Europa. ha riferito in merito alle misure precauzionali adottate dal Messico e dagli Stati Uniti e che assumeranno via via tutti i Paesi che registreranno casi di contagio.

siamo in quella fase in cui c'è trasmissione da uomo a uomo, con la possibilità di scatenare focolai endemici. A tale proposito, è importante capire anche lo stato del Piano pandemico nazionale: che il Ministero abbia adottato da tempo tale piano anche in base alle direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità è un fatto importante; il Ministero tuttavia non ha una visione globale dei piani pandemici, come il ministro Sacconi ha testé evidenziato (la riunione si svolgerà domani). Quindi, non so se è in grado di dirci se tutte le Regioni hanno un piano pandemico e sono in grado di attuarlo. mondiale della sanità, il Piano pandemico nazionale prevede una messa a punto di piani di emergenza per mantenere i servizi sanitari e gli altri servizi essenziali.

si riproponga la necessità di ripristinarlo; una misura che non può essere più rinviata se si ha a cuore la salute dei cittadini. dei cittadini. Il Ministero del welfare, a questo punto, in accordo con i Dicasteri coinvolti, deve identificare il personale che può essere mobilitato e coinvolto per fornire assistenza sanitaria in caso di pandemia e sviluppare una lista di servizi essenziali. Per ognuno dei servizi essenziali individuati deve identificare il responsabile e mettere a punto i piani di emergenza che includano le procedure per coprire le assenze durante la pandemia. Per ogni servizio essenziale deve compilare ed elencare un numero di persone, la cui assenza pone in serio pericolo la sicurezza ed interferisce pesantemente con la risposta alla pandemia. pandemia. Il Piano pandemico nazionale, inoltre, prevede un piano di formazione per gli operatori in modo da sviluppare le conoscenze sulla pandemia per essere capaci di interventi pronti e appropriati. Sono previste, per esempio, simulazioni ed esercitazioni, che sono obbligatorie. Siamo in grado oggi di fornire tutte queste cose che sono previste nel Piano pandemico nazionale? Siamo in grado di offrirle su tutto il territorio nazionale?

seguire? I primi presidi territoriali, per esempio le farmacie, hanno a disposizione tutte le notizie necessarie, sia per reperire i farmaci disponibili che per fornire le

Ci fa ben sperare l'immediata risposta delle industrie farmaceutiche che, secondo quanto riferito da Farmindustria, stanno già lavorando al vaccino contro l'influenza suina. Come sappiamo, i tempi non saranno brevi e ci vorranno dei mesi. dei mesi. Credo che sia decisivo anche il ruolo internazionale. Chiedo in che misura il Governo stia contribuendo, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Unione europea, alla formazione di una posizione e di una strategia comune per il contrasto e la prevenzione dell'influenza suina. infine, che serva una giusta comunicazione sociale, che sia soprattutto in grado di dirci come stanno realmente le cose e di evitare anche un'irrazionale psicosi, che può sicuramente danneggiare l'organizzazione sanitaria e le strutture che devono, invece, operare in modo sereno e proporzionato. Ritengo che su questo - sono d'accordo con lei - ci sia la necessità di un corretto atteggiamento sotto il profilo sanitario e le chiedo, anche a nome della Commissione

signor Ministro, signor Sottosegretario, dopo tante informazioni non controllate finalmente oggi abbiamo sentito in quest'Aula alcuni punti chiari. non si trasmette con gli alimenti (ancora oggi sono arrivate numerosissime telefonate al numero verde che il Ministero ha istituito da parte della popolazione che chiede come bisogna regolarsi con gli alimenti); si trasmette da uomo a uomo per via aerea, ed è su questo che dobbiamo lavorare. presente in forma endemica in Messico, è presente negli Stati Uniti e credo che si vada affacciando anche in Europa. Tuttavia, in Italia al momento - lo sottolineava il Ministro qualche minuto fa - abbiamo avuto la capacità di intercettare 11 casi sospetti, ma nessuno di questi si è dimostrato reale. Che cosa ci deve preoccupare realmente? Da una parte, come prevenire tutto questo e come evitare il contagio; dall'altra, cercare di affrontare l'eventuale presenza qualora questa dovesse intervenire.

agli aeroporti, ai porti, con una rete di collegamento tra i medici di medicina generale e i laboratori dedicati all'identificazione in tempi molto rapidi. In questo vorrei tranquillizzare la collega Bianchi, perché il sistema di controllo tra i medici di medicina generale e i laboratori dedicati è estremamente rapido e in ventiquattr'ore è possibile ottenere la risposta adatta. Costante è il funzionamento del centro controllo delle malattie gestito dall'Istituto superiore di sanità.

un costante controllo d'intesa con le Regioni. Nella mia regione ho potuto constatare ieri come ci sia già un'organizzazione preposta a verificare eventuali casi. Ed è lì, soprattutto nelle regioni, che bisogna lavorare con un controllo primario.

Diciamo con chiarezza no ad allarmismi inutili e dannosi. Ancor oggi agenzie di stampa fomentavano inutili allarmi: incapacità, insufficienza degli interventi, quando abbiamo verificato e sentito oggi che ciò non è assolutamente vero. un richiamo, indipendentemente dalla componente politica, perché in queste situazioni vi sia un comportamento sempre più responsabile: non creiamo panico, aiutiamo informazioni esatte. Anche l'Unione europea invita a non diffondere panico. Mi permetto di invitare il Ministro a preoccuparsi in tempi rapidi di completare la nostra dotazione di farmaci e di abbinare con l'Unione europea la valutazione dell'opportunità della proclamazione dell'intervento vaccinale. Domani è già previsto un'incontro della Commissaria alla sanità europea con le aziende. Le scelte in questo settore e le scelte nel campo vaccinale non possono essere dedicate ad una realtà territoriale: la scelta sanitaria di un Paese incide sui rischi degli altri. Dobbiamo necessariamente ragionare insieme con l'Unione europea per giungere a valutazioni e conclusioni univoche. Non abbassiamo la guardia. iniziative di maggior controllo alle frontiere e ai sistemi regionali, con particolare attenzione all'efficacia dei reparti di malattie infettive; una massima attenzione all'informazione per fronteggiare inutili e negativi allarmismi.

in particolare Valchiusella, Cervo, Sesia, Orco, Lanzo e Sangone, oltre che una parte del bacino del Toce. Con questo intervento voglio fare una segnalazione all'Aula, nonché un invito al Governo a prendere in immediata considerazione la richiesta urgente, inviata dalla Regione Piemonte, di proclamare lo stato d'emergenza e ottenere immediatamente gli strumenti per poter intervenire.

Signora Presidente, nella relazione scritta do conto delle modifiche che il disegno di legge sul federalismo fiscale ha subito durante l'*iter* alla Camera dei deputati.

le modifiche sono state importanti e significative, ma l'impianto e gli assi portanti del disegno di legge sono stati confermati anche dall'altro ramo del Parlamento.

Innanzitutto va detto che il testo approvato è frutto di un intenso lavoro svolto sia dalle forze della maggioranza, sia da quelle dell'opposizione, e naturalmente anche da parte del Governo. L'opposizione, com'è noto, ha contribuito alla definizione dei contenuti del provvedimento mediante proposte emendative che presso ciascun ramo del Parlamento hanno trovato accoglimento da parte del Governo. Tuttavia, vi sono alcuni temi sui quali l'opposizione ha manifestato ancora un'insoddisfazione anche nel corso dell'esame in terza lettura da parte delle Commissioni riunite, presentando pertanto appositi emendamenti. Lo stato del dibattito, il livello di condivisione del testo - che è frutto, lo ripeto, di un intenso lavoro sia durante il passaggio al Senato che durante quello alla Camera - e l'economia complessiva dei lavori non hanno consentito di approvare ulteriori emendamenti; ma ciò non esclude, rende anzi auspicabile, che su tali argomenti possa esservi lo spazio per ulteriori approfondimenti. In tal senso il Governo ha già manifestato la disponibilità a valutare con attenzione gli eventuali ordini del giorno che l'opposizione dovesse presentare durante questa terza lettura. Senza elencare dettagliatamente tutte le singole tematiche rimaste per così dire aperte, giova dare conto di alcune. Si tratta, in primo luogo, del tema della Carta delle autonomie locali, un punto che dovrebbe costituire indubbiamente la partenza per una definizione degli assetti delle competenze degli enti locali, al fine della successiva individuazione dei livelli di finanziamento.

sui tempi per la presentazione in Parlamento del testo della Carta delle autonomie locali, tanto che la stessa opposizione ha manifestato soddisfazione per la puntualità

oggetto di particolare attenzione, è quello relativo al Patto di stabilità interno. In relazione ad esso è stata evidenziata la difficoltà attuale, data dal fatto che molte gestioni di bilancio degli enti locali risultano altamente a rischio di mancato rispetto dei vincoli del Patto di stabilità, in particolare in relazione alle spese per opere infrastrutturali già deliberate ed assegnate con procedura di affidamento ed in corso di esecuzione.

Come è noto, l'opposizione ha chiesto di introdurre queste tematiche nel novero dei livelli essenziali delle prestazioni vi sono state proposte emendative da parte dell'opposizione tendenti ad un ritorno al testo approvato dal Senato in prima lettura.

Un'altra questione aperta è rappresentata poi dal tema della migliore definizione dei fondi perequativi, nonché del mancato inserimento dei beni culturali e dell'edilizia scolastica tra le funzioni fondamentali. Anche questo tema è stato più volte oggetto di discussione; si sono fatti passi in avanti rispetto al testo che prima il Senato e poi la Camera hanno approvato, ma l'opposizione ha ritenuto di dover presentare anche in questo caso proposte di carattere emendativo.

qui comincia il compito impegnativo di elaborazione e stesura dei decreti delegati; ma siamo pronti a questo, convinti che

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, ciascun Gruppo di opposizione valuterà alla fine dei lavori quale giudizio dare dei provvedimenti in esame, anche alla luce delle disponibilità di Governo e maggioranza ad accogliere ulteriori proposte in termini di emendamenti ed ordini del giorno. E ciascuno lo farà sulla base delle proprie specifiche motivazioni. Il Gruppo del Partito Democratico, principale Gruppo di opposizione, ha già espresso, durante i lavori delle Commissioni riunite, un giudizio positivo sulle modifiche intervenute nel corso del dibattito parlamentare al disegno di legge oggi al nostro esame. Queste modifiche non sono ancora sufficienti per disporre di un testo nel quale il PD possa pienamente riconoscersi.

verso una legge condivisa su di un tema molto rilevante come il federalismo fiscale. Il Governo, con il ministro Roberto Calderoli, e la maggioranza, con il relatore Antonio Azzollini, durante la prima lettura del provvedimento hanno condotto la discussione con uno spirito di apertura autentica al confronto con le proposte provenienti dall'opposizione. È importante che questo spirito non venga meno proprio ora, poiché ci sono alcune questioni molto rilevanti che devono essere ancora affrontate. Da come esse verranno risolte dipenderà il giudizio su un punto per noi fondamentale, cioè se si vuole aprire davvero una fase di cambiamento in senso autonomista e federalista della nostra Repubblica oppure se ci si vuole limitare ad uno *spot* elettorale. Quando si discute di questioni attinenti alla Costituzione e alla sua attuazione, nonché alle fondamentali regole del gioco democratico, la ricerca di soluzioni condivise non dovrebbe mai venire meno. Questa, in ogni caso, è la ferma intenzione dell'opposizione che vuole distinguere costantemente il piano della battaglia politica e parlamentare da quello della ricerca dell'intesa sulle regole. È doveroso ricordare che in almeno due occasioni, entrambe successive all'approvazione in prima lettura del disegno di legge sul federalismo fiscale da parte del Senato, Governo e maggioranza non si sono comportati in questo modo. Mi riferisco all'uso della decretazione di urgenza sul caso Englaro e alla fissazione della data per il *referendum* elettorale, a parte una parziale intesa raggiunta proprio oggi in Commissione affari costituzionali, che noi stessi abbiamo ritenuto essere il male minore e non la soluzione ottimale. Non ci possono essere due pesi e due misure in materia di applicazione della Costituzione e di regole della democrazia. Non può esserci la ricerca dell'intesa solo sui temi che interessano la maggioranza, o una parte di essa, per poi procedere unilateralmente su tutto il resto. saremo fermi nel denunciare questi comportamenti ma saremo anche pronti a riconoscere la reale volontà di procedere insieme, come avvenuto nella prima discussione in Senato sul federalismo fiscale e come ci auguriamo che possa avvenire anche ora. ora. Siamo fermamente interessati all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il Partito Democratico ha creduto fin dall'inizio nella bontà del nuovo Titolo V, il quale su qualche punto potrebbe certamente essere migliorato. si riconosce in pieno nell'esigenza di attuare il federalismo previsto dalla Costituzione. Se non fosse stato così - sia chiaro sia il PD che l'Italia dei Valori non avrebbero deciso di contribuire positivamente all'elaborazione della legge oggi al nostro esame, esponendosi alla critica di lasciare che la Lega Nord potesse sventolare la sua bandiera in vista delle prossime elezioni amministrative. L'UDC, come è noto, ha fatto una scelta diversa, che motiverà durante la discussione in Aula. Noi siamo convinti di aver contribuito in modo determinante a migliorare il testo del disegno di legge. Se vi è una bandiera da sventolare ora, è quella del federalismo cooperativo voluto dalla nostra Costituzione e non quello del modello lombardo presentato in campagna elettorale dall'alleanza tra Popolo delle Libertà e Lega Nord, di cui non vi è più alcuna traccia nel testo che stiamo discutendo. Dalla risposta che darete ai nostri interrogativi, contenuti negli ordini del giorno che presenteremo, dipenderà non solo il nostro giudizio ma l'indirizzo che prevarrà anche al vostro interno nell'attuazione della legge. È innegabile, infatti, che vi siano orientamenti diversi anche all'interno della maggioranza. Le dichiarazioni di ieri del ministro dell'economia Giulio Tremonti, secondo il quale le riforme non si fanno in tempo di crisi, a mio modo di vedere dovrebbero preoccupare anche i Ministri della Lega Nord. È evidente infatti che, in questo modo, il ministro Tremonti ribadisce un giudizio, da lui chiaramente espresso con le sue ripetute assenze in questa discussione, secondo il quale su tutta questa materia il Ministero dell'economia si riserva di dire la sua opinione a tempo debito.

Per questo motivo è molto importante, come propone di fare il PD con i quattro ordini del giorno che abbiamo presentato, chiarire le condizioni di contesto in cui si colloca la discussione sulla legge che ora è al nostro esame. Il federalismo fiscale non può essere come la tela di Penelope, con qualcuno nel Governo che disfa di notte quello che altri fanno di giorno. Mentre si predica il federalismo fiscale non si può praticare un centralismo esasperato che soffoca gli enti locali. Non si può ritardare ancora il cammino parlamentare della Carta delle autonomie locali. Non si possono negare le simulazioni circa la redistribuzione territoriale delle risorse prodotta dal provvedimento. Non si può rinviare ancora l' *iter* legislativo per una modifica costituzionale che introduca una Camera delle autonomie in sostituzione dell'attuale Senato e differenzi le sue funzioni rispetto all'altra Camera. Vi sono quindi molte ragioni per ritenere che questa discussione non è assolutamente inutile. Non è un passaggio burocratico, ma è il momento nel quale possiamo verificare chi vuole far sul serio e chi no. Comincio con l'illustrare l'ordine del giorno G101, relativo al Patto di stabilità interno per gli enti locali, che ha come prima firmataria la presidente del nostro Gruppo Anna Finocchiaro.

che prevedeva impegni molto precisi e stringenti, come ad esempio la compensazione dovuta agli enti locali per la perdita del gettito ICI sull'abitazione principale e modifiche al Patto di stabilità interno per rendere possibile l'impiego delle risorse che Comuni e Province hanno soprattutto per gli investimenti.

con il risultato di una crisi gravissima che si ripercuote sul settore dell'edilizia. L'associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha calcolato in 130.000 il numero di posti di lavoro persi in questo settore strategico a partire dall'inizio della crisi. cosa si aspetti ad intervenire con decisione per consentire ai Comuni e alle Province di impiegare queste risorse per favorire gli investimenti. Alla Camera, qualche giorno dopo l'approvazione di quella mozione, il Governo ha presentato una norma nel decreto anticrisi, poi riproposta anche qui al Senato con il ricorso al voto di fiducia, che va in direzione opposta rispetto alla Con l'ordine del giorno Finocchiaro proponiamo di nuovo alla maggioranza e al Governo di rispettare gli impegni contenuti nella mozione Franceschini, ma aggiungiamo un elemento molto importante: qualora entro il mese di giugno non ci sia una nuova normativa sul Patto di stabilità interno, proponiamo di abolire le sanzioni per i Comuni e le Province che sono costrette a non rispettare il Patto per pagare investimenti già decisi. Vi è una situazione urgente di crisi economica che motiva un provvedimento di questa natura.

il Governo, perché non ha rispettato l'impegno assunto in quest'Aula di presentare la Carta delle autonomie locali a poche settimane di distanza dal voto sul federalismo fiscale in Senato. Il Governo ha presentato un nuovo impianto, che abbiamo riconosciuto essere più innovativo rispetto a quello precedente, anche perché in questo caso il Governo si è ampiamente ispirato al testo presentato dal Partito Democratico.

all'unificazione degli uffici periferici dei Ministeri centrali negli uffici territoriali del Governo. Per noi questo è un punto fondamentale, perché da lì si può ottenere un nuovo trasferimento di funzioni verso il sistema delle autonomie locali. Si possono ottenere una razionalizzazione, uno snellimento ed anche una riduzione dei costi.

e la difesa che avevamo escluso anche noi. Se si adottasse questa soluzione si ridurrebbe esattamente della metà l'impatto positivo di una norma del genere. Quindi, invitiamo il Governo a spingersi oltre, ad essere più coraggioso, Il terzo ordine al giorno, il G104, si riferisce al complesso delle riforme istituzionali e costituzionali necessarie per sostenere il federalismo fiscale.

Per poterlo fare è necessario differenziare le funzioni, ridurre il numero dei parlamentari e trovare un nuovo equilibrio tra il potere legislativo ed il potere esecutivo nell'ambito della forma di governo parlamentare prevista dalla nostra Costituzione. Questo ordine del giorno che ha come primo firmatario il vicepresidente vicario del nostro Gruppo, senatore Luigi Zanda, propone, come è accaduto alla Camera, di ripartire dalla bozza Violante.

prodotti nella distribuzione territoriale delle risorse dalla legge che stiamo per approvare; questione che i colleghi conoscono bene e su cui noi abbiamo insistito moltissimo. Sappiamo quello che ci ha detto il quest'Aula il ministro Tremonti: non è possibile conoscere il risultato finale del processo, perché manca ancora la valutazione dei costi standard che devono sostituire la spesa storica. Ma quel che chiediamo è ciò che è perfettamente possibile e che molti istituti universitari già stanno facendo: le simulazioni circa gli effetti redistributivi del provvedimento. Se finora ciò non è accaduto, abbiamo ragione di pensare che il Governo e la maggioranza non hanno voluto,

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, nella relazione scritta vedrete una serie di osservazioni puntuali circa le modifiche intervenute e i punti che riteniamo ancora aperti. aperti. Intendo qui enunciare solo le questioni fondamentali. Ci sono tre grandi modifiche, frutto del contributo dato principalmente dal Gruppo del Partito Democratico e che rivendichiamo come utili e positive per il Paese. La prima riguarda la Commissione parlamentare che consentirà un controllo effettivo sulla delega affidata al Governo. La seconda è l'introduzione del Patto di convergenza per consentire ai territori meno dotati di servizi di adeguarsi

che dovrebbero verificare la congruità delle risorse attribuite fin dal momento successivo all'approvazione degli Statuti, cioè dal 1948. Questo ci sembra eccessivo, mentre ci sembra invece più utile e congruo tornare al testo approvato dal Senato. riguarda l'elencazione delle Città metropolitane: l'aver introdotto la città di Reggio Calabria è un'evidente forzatura che con il tempo pagheremo, perché ci saranno pressioni da parte di altre città per entrare in quell'elenco, che se sarà così non avrà più significato.

Restano altri punti, su cui peraltro correttamente il collega Azzollini prima è intervenuto, che comunque ci fanno esprimere un giudizio non

comporterebbe una nuova lettura, ma secondo noi sarebbe la condizione per arrivare ad un testo pienamente condiviso. In ogni caso, sia chiaro, il nostro atteggiamento, e lo ha dimostrato il comportamento che abbiamo assunto nelle Aule parlamentari, non è minimamente dovuto

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è difficile che, prendendo la parola, si debba riconoscere, come sto per fare

come ben sappiamo - alla revisione di alcuni degli assetti organizzativi in materia fiscale, in una logica solidaristica del nostro Paese. Il collega Vitali, sia nel merito che nel metodo, con grande onestà intellettuale, pur evidenziando una ancora non sufficiente convergenza, al punto da portare il Partito Democratico ad una valutazione positiva e quindi all'espressione di un voto favorevole, esprime un apprezzamento per i metodi ed il merito del provvedimento in esame. Vorrei ringraziare in proposito, oltre che il presidente Azzollini, per la consueta abilità e

il Ministro per le riforme, per l'equilibrio e l'apertura con i quali ha saputo dare ascolto alle istanze di tutte le parti istituzionali e politiche, confrontandosi con loro senza rigidità pregiudiziali e accogliendo ogni contributo utile a migliorare il testo del disegno di legge delega. È stato, infatti, poc'anzi ricordato che il testo, oggi in seconda lettura

approvati con una manciata di voti e con grosse perplessità. Un ringraziamento permettetemi di rivolgerlo anche ai colleghi deputati che, proseguendo nel solco del lavoro condotto da quest'Aula, nell'altro ramo del Parlamento hanno saputo apportare al testo del disegno di legge importanti modifiche che hanno prodotto il risultato di ridurre ulteriormente le contrapposizioni su una riforma che non può essere considerata di una parte sola, ma di tutto il Paese, quale che sia la parte politica o la Regione cui appartengono. Il lavoro congiunto di Senato e Camera credo sia la risposta migliore alle Cassandre che un giorno si e l'altro pure annunciano la fine del Parlamento e della sua funzione legislativa. le Assemblee legislative hanno invece dimostrato che in queste Aule le leggi si formano attraverso un confronto serio,

nel vivo della riforma, non tanto per ripercorrerne i contenuti, noti a voi tutti, quanto per rispondere a chi, *vox clamantis* nel deserto del suo isolamento politico, ha ritenuto anche alla Camera dei deputati di definire questa riforma come una riforma *slogan,* una riforma che non c'è. Bene, vorrei dire a chi l'ha bollata come tale che, se questa riforma è un fantasma, io, che ai fantasmi non ho mai creduto, comincerò a crederci forse proprio da adesso perché in effetti, come ogni fantasma che si rispetti, questa riforma produce un rumore di catene, ma è rumore di catene finalmente spezzate, non trascinate. E non mi riferisco alle catene care all'iconografia degli amici della Lega, quelle che manterrebbero il Nord assoggettato al centralismo romano, a ceppi di ben più concreto peso storico, quelli rappresentati dall'inerzia di quella classe politica che ha mancato di avviare sin qui la fase di riforme che il Paese attende anche per avviare un serio processo di modernizzazione. Altro che fantasma, cari colleghi: questa è una riforma dall'architettura solida, resa ancora più convincente dal decisivo

al Senato. Una di queste riguarda la riserva d'aliquota IRPEF per le Regioni, che viene abolita e sostituita come fonte di finanziamento per le funzioni essenziali con compartecipazioni

tavoli di confronto singoli tra il Governo e ciascuna Regione per definire il concorso delle autonomie speciali alla perequazione. altro passaggio rilevantissimo che rappresenta un passo in avanti nell'architettura di questo importante provvedimento si riferisce alle funzioni della cosiddetta bicameralina sui decreti attuativi, che vede il suo ruolo ulteriormente rinforzato: la Commissione, infatti, non soltanto avrà una funzione di controllo, ma anche di indirizzo. Sono state rafforzate anche le norme che disciplinano la perequazione verticale per assicurare i livelli di assistenza essenziali,

alla piena attuazione degli articoli della Costituzione - il 29, il 30 e il 31 - inerenti ai diritti della famiglia. Credo però che la chiave di volta del provvedimento provvedimento resti il superamento del criterio della spesa storica, fonte perenne di sperequazioni, soprattutto a danno del Sud. Con la riforma, per ogni servizio erogato dagli enti territoriali si individuerà un «costo *standard*», al quale tutti dovranno uniformarsi durante un periodo transitorio di cinque anni. Si eliminerà così il meccanismo perverso che finora, facendo riferimento alle spese pregresse, premiava con maggiori risorse gli enti che spendevano di più, e si introdurranno al tempo stesso condizioni di maggiore trasparenza nella gestione della spesa per salute, istruzione e servizi sociali, eliminando le improduttività, le sacche di inefficienza, l'assistenza che finisce per diventare un opaco assistenzialismo in cui hanno modo di prosperare più facilmente il malcostume e la corruzione. È una riforma realista e prudente, signor Ministro, che sa che per una svolta così radicale occorrono tempo, cautela ed un monitoraggio continuo durante l'applicazione: gli strumenti previsti dalla legge agli articoli 3, 4 e 5, con le due Commissioni e ampie garanzie, sia per una traduzione in atti del provvedimento, coerente con i principi di equità, efficienza e logica solidale che lo ispirano, sia per il rispetto di due principi fondamentali della Costituzione: quello dell'uguaglianza e quello della buona amministrazione. È una riforma, infine, che rappresenta l'inizio di un percorso che dovrà sfociare in una più larga revisione degli assetti istituzionali dello Stato. Il federalismo fiscale, che rafforza il momento periferico, infatti, impone coerenti e conseguenti interventi di bilanciamento a livello centrale, sia sull'Esecutivo sia sull'Assemblea legislativa, che devono essere entrambi posti in condizione di esercitare i loro poteri con efficacia reale. Ma queste sono le esaltanti sfide che il Parlamento, insieme al Governo, sarà chiamato ad affrontare domani. L'oggi si chiama federalismo fiscale,

la parte d'Italia dove, con malizia strumentale, la riforma federalista è stata spesso presentata come un attentato agli interessi del Meridione. Sono convinto dell'esatto opposto: le condizioni di difficoltà delle Regioni del Sud possono essere superate soltanto con uno scatto in avanti che - prima e più che economico - è culturale, politico e sociale. il ritardo di sviluppo del Sud non è una causa, ma il prodotto del *deficit* di cultura politica di una classe dirigente che, dimenticando l'orgoglio della propria storia, non ha saputo e forse non ha voluto tutelare in maniera adeguata la libertà, l'autonomia e la dignità

in una logica di proiezione verso lo sviluppo. Questo federalismo fiscale, dunque, non è nemico del Sud: i nemici veri sono gli idolatri dell'immobilismo, quelli che ai meccanismi rugginosi della macchina amministrativa attuale non vogliono rinunziare, non perché funzionali agli interessi del Mezzogiorno, ma perché permettono loro di tutelare i propri. è anche e soprattutto, per il Sud, un'opportunità, una scelta di progresso, che produrrà un nuovo modo di pensare ed una classe dirigente che dovrà combattere in prima fila - pena la perdita del consenso la guerra alle inefficienze, agli sprechi, alla corruzione di ogni tipo, guadagnandosi la credibilità necessaria a rivendicare i diritti del Mezzogiorno, con la testa alta e con le carte in regola, perché un Mezzogiorno nuovo

Quella lezione è sempre attuale, per il Sud, come per il Centro, come per il Nord, in una logica di unità nazionale ed è una lezione che è ben presente nel disegno di legge delega sul federalismo che lancia con coraggio un'autentica sfida di modernità e responsabilità a tutti gli italiani. Essa è una sfida che tutela gli amministrati e responsabilizza gli amministratori, che ricongiunge l'onere della spesa con l'onere della tassazione; una sfida che bisogna ora raccogliere e portare avanti con concretezza, perché questa legge è una delle porte attraverso le quali passa il futuro del Paese. Una porta, signora Presidente (e la ringrazio per il tempo supplementare concessomi), che abbiamo il dovere di varcare con prudenza, con equilibrio e senza alcun indugio.

siamo ad un anno dall'insediamento del Senato e dall'avvio della XVI legislatura e credo ci sia soddisfazione nella maggioranza, nella Lega in particolare, per aver portato a buon fine il provvedimento di delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Non era né ovvio, né scontato. È stato un anno di crisi ed è oggi un tempo di crisi; crisi globale, crisi della quale nessuno sa dire quanto durerà, come evolverà. Gli analisti economici ci dicono che la portata della crisi attuale è superiore a quella del 1929, anche se per fortuna le conseguenze sociali saranno più contenute, soprattutto perché la dimensione della finanza pubblica è oggi molto superiore a quella del secolo scorso e rappresenta una garanzia di spesa e di sostegno della domanda. Tuttavia, pur escludendo le catastrofi sociali del secolo scorso, è sicuro che gli effetti della crisi saranno ancora molto gravi e particolarmente dolorosi proprio per le situazioni e le persone socialmente più deboli. Ovunque la crisi sta creando problemi sociali rilevanti, ma la cifra di questa crisi, la parola chiave, è fiducia, o meglio la diffusione di un clima generale di sfiducia nelle classi dirigenti. Quello che viene in luce qui, nel nostro Paese, anche se per la verità il Governo fa di tutto per oscurarlo, è che c'è una scala di valori, su cui si è fondato il nostro modello di crescita, che oggi non è più accettabile, perché proprio di fronte ad una crisi con queste caratteristiche generali si dimostra che il sistema è incapace di assicurare livelli civili di sicurezza sociale e di solidarietà. Solidarietà: questa parola tanto bistrattata, e non solo da destra, in momenti come questo assurge a tutto il suo valore di parola chiave, cardine, priorità nell'organizzazione della vita civile e per la politica. Sono purtroppo le famiglie più giovani, quelle che dovrebbero essere il nerbo della costruzione del futuro del nostro Paese, ad essere spesso le più colpite, perché i primi a pagare sono i lavoratori precari e le giovani donne. Trovarsi poveri può succedere in un momento: con la cassa integrazione per lui, la perdita di un contratto a tempo determinato per lei, il mutuo e la retta dell'asilo E in Italia, oltre che poveri, ci si sente abbandonati; abbandonati da uno Stato che si dimostra incapace di intervenire, da una politica che si occupa molto di simboli, di *media*, di ricreazione del popolo, ma in realtà non presta alcuna attenzione ai bisogni del sociale e alla vita delle persone. Proprio dentro questa crisi e in questo anno gli italiani hanno potuto e possono toccare con mano quanto siano diseguali tra loro e portatrici di ulteriori diseguaglianze le misure di sostegno dei redditi. E anche noi, qui, dobbiamo dirci la verità: abbiamo verificato un fatto molto triste, cioè che mentre sul federalismo fiscale dobbiamo promettere e impegnarci a garantire solidarietà tra le Regioni più ricche e quelle più povere e questo tutti abbiamo provato a fare, in pratica quel che è accaduto nel Paese è esattamente il contrario. Infatti, si calcola che le risorse destinate al Sud, corrispondenti ad un punto di prodotto interno lordo, siano state dirottate a beneficio del Nord o comunque di obiettivi di interesse generale.

di come Nord e Sud siano bensì diversi, ma anche molto simili; di come sfiducia ed incertezza si siano diffuse a tutte le latitudini; di come spesso in Italia chiamiamo «Mezzogiorno» tutto quello che non ci piace, che non vogliamo vedere del nostro Paese (come le mafie, ad esempio) o i problemi difficili che non riusciamo a risolvere, mentre non è così. Risolvere i problemi del Mezzogiorno e i problemi dell'Italia richiede la stessa strategia di fondo, richiede di elaborare una strategia. Questo spetta alla politica, ma a quale politica? Quella di una Lega del Sud contro la Lega Nord? Penso che la politica di cui abbiamo bisogno come Paese non è quella di anteporre sistematicamente grazie futuro e richiede lo stesso coraggio che ebbero i nostri Padri costituenti, che provarono a costruire quel Paese, quella società, che ancora oggi noi non abbiamo; siamo ancora molto lontani da tutto ciò, anche se quest'anno abbiamo lavorato a tal fine. Per questo, questo, l'esito parlamentare della delega sul federalismo fiscale risulta o può risultare astratto, avulso dal Paese reale. reale. In questo momento, sentiamo crescere i rischi legati al disagio sociale e all'aumento delle disuguaglianze, delle sperequazioni tra aree del Paese e tra gruppi sociali, tra generi e generazioni, più che in tutti gli altri Paesi europei. In qualità di senatrice eletta nel Mezzogiorno, mi sono avvicinata al dibattito sul federalismo con molte attese e preoccupazioni. Le preoccupazioni e i rischi sono evidenti. Sul piano generale, vi è il rischio fondato ed ampiamente discusso che vede una relazione tra le iniziative di devoluzione e l'aumento delle disuguaglianze, ma anche fatti più concreti: la base di redditi cui applicare le tasse e i contributi locali nel Mezzogiorno è più limitata, perché il reddito per abitante è poco più della metà di quello del Nord e perché è molto più estesa l'economia irregolare. Le attese e le potenzialità invece riguardano la responsabilità degli amministratori nel rapporto con i cittadini e questo rimanda alla qualità dell'amministrazione, dei servizi, alla trasparenza, all'innovazione necessaria, cimento e percorso sfidante per il buon governo. Ai problemi gravi che il tema solleva nel rapporto con la pubblica amministrazione meridionale la proposta che abbiamo elaborato è stata via via capace di individuare soluzioni credibili.

anche se a molti problemi francamente oggi io non saprei rispondere con certezza: se cioè la perequazione sarà sufficiente a garantire ai cittadini del Sud i servizi fondamentali; se i costi standard della sanità dei trasporti locali possano effettivamente stimolare il buon governo locale. Ovviamente non tutte le risposte si possono avere in questo momento; è certo, però, che il federalismo fiscale, per evitare conseguenze rovinose nel Sud, deve reggersi su due pilastri: il buon governo locale della pubblica amministrazione e la solidarietà prestata da tutto il resto del Paese. In questo senso, resta ancora molto da fare, anche se la Camera dei deputati, accogliendo diversi emendamenti presentati dall'istituto SVIMEZ, ci rimanda un testo che al Sud dà qualche

"bagnato nelle acque" di un confronto politico che ha permesso all'opposizione di esprimere importanti suggerimenti, molti dei quali anche accolti. Pertanto, oggi abbiamo di fronte una soluzione conclusiva che appare sicuramente più equilibrata. Abbiamo di fronte soprattutto una questione: noi ragioniamo attorno a un disegno di legge, che è l'attuazione dell'articolo 119 del Titolo V. V. Attorno al Titolo V la riflessione, a mio giudizio, andava svolta forse con più serenità e approfondimento. È vero che ci consegna un'indicazione robusta molto coraggiosa, ma apre anche dei problemi: l'aver cancellato il pilastro dei trasferimenti, averlo considerato come un impaccio e un elemento negativo e aver esaltato, di converso, il ruolo, la funzione e il primato assoluto dell'autonomia impositiva e tributaria crea un nuovo equilibrio molto più problematico di quello che noi usualmente abbiamo detto anche nei nostri lavori di Camera e Senato. In realtà, avendo cancellato un tipo di ordinamento che aveva nei trasferimenti la leva di forza per realizzare un equilibrio tra diversi Comuni, Province e Regioni, con la possibilità di una manovra organica che garantisse quasi immediatamente il primo livello e quello conclusivamente più organico della perequazione, oggi noi siamo costretti ad agire con molto più affanno, più perizia, con tutta una serie di cautele, di misure e, secondo me, con un sovraccarico di questioni che sopraggiungeranno fatalmente. Ha ragione, a mio giudizio, il professor Giarda quando dice che, pensando di creare un ordinamento tutto nuovo, stiamo tornando all'ordinamento della finanza locale del 1931 che, a sua volta, era tributaria della riforma vigente subito dopo l'unità d'Italia.

l'imposizione sugli immobili è la vera competenza dei Comuni; quindi, si dice che questo è il nuovo orizzonte. Ma è un orizzonte che già esiste, perché già oggi i Comuni hanno in mano la leva dell'ICI. Il Governo e la maggioranza però non ci dicono se, ad esempio, un un domani rimarrà il regime - sto parlando di quello che conosciamo da qualche mese a questa parte - dell'imposizione sugli immobili che grava su tutti i cittadini, meno che su quelli proprietari dell'abitazione principale. A questo punto ci sarebbe da domandarsi come sia possibile, anche da un punto di vista strettamente costituzionale, che tutti i servizi debbano essere sostenuti finanziariamente da tutti i cittadini, che in questo caso, visto che i proprietari di prima casa sono esonerati da questa imposta, che appunto dovrebbe servire a finanziare le attività e le funzioni amministrative locali. Credo che dobbiamo essere più puntuali e più attenti e che non dovremmo farci prendere dall'entusiasmo. Ecco perché l'astensione del Partito Democratico va presa molto sul serio. Dalla Camera ci torna un testo che haqualche amenità. lo dico al ministro Bossi - non so francamente da dove sia stato possibile ricavare (conosco il dibattito politico e scientifico di questi ultimi venti anni, sia pure sommariamente) che Reggio Calabria è una città metropolitana.

quello che oggi è il Consiglio comunale non sarà più tale? È una cosa abbastanza misteriosa.

sull'imposta sul reddito, che avrebbe generato tanti regimi diversi per il nostro ordinamento fiscale: tante Regioni, altrettanti diversi ordinamenti fiscali. Fra le molte incognite

ma questa è una scorciatoia. Non mi dilungo, ma si tratta - ripeto - di una scorciatoia sulla quale il Partito Democratico non è d'accordo perché il presidenzialismo - l'abbiamo ripetuto più volte è una risposta sbagliata ad un'esigenza giusta. L'esigenza giusta è la governabilità, la razionalità del sistema, la risposta sbagliata è quando, utilizzando il presidenzialismo, si personalizza ancor di più la politica, la si centralizza e la si verticalizza. Sarebbe un errore e noi oggi, discutendo di federalismo fiscale e guardando avanti, dobbiamo dire che questo errore non dobbiamo compierlo. *(Applausi

nell'esistenza personale, come nella storia dei popoli, si presenta il momento in cui gli uomini di buona volontà sono chiamati a far appello alle proprie doti di coraggio e fiducia nell'avvenire, per cambiare ciò che, sino a non molto tempo prima, appariva nell'opinione comune immutabile ed insostituibile. Ben di rado accade, in simili frangenti, che il nuovo cammino si offra già tracciato e sicuro a chi vi accede. Il più delle volte, ogni grande cambiamento s'accompagna ad ostacoli e travagli, ma quando scocca l'ora del rinnovamento, quanti rimangono in prudente attesa ne restano travolti, al pari di chi vi si oppone. Coloro che, invece, confidano nella giustezza delle proprie convinzioni e nella consapevolezza che il momento atteso è giunto, sperimentano quella condizione creativa di Stato nascente e s'impegnano anche in assenza di confortanti garanzie assolute, poiché ogni remora viene superata in loro dalla forza del maturato convincimento. E siccome resto persuaso che un'ampia maggioranza di colleghi parlamentari abbia innegabilmente acquisito un sincero e genuino orientamento federalista, mi rincresce avvertire in certe prese di posizione le briglie tese della ritrosia, il morso del freno inibitorio, l'ancestrale paura d'infrangere il tabù: di cosa si alimenta, altrimenti, questa titubanza che induce alcuni dell'opposizione a pretendere nero su bianco cambiali, in pegno, al più, d'una timida astensione? Oggi dovremmo riferirci allo Statuto Albertino, se i Costituenti avessero condizionato il proprio assenso alla preventiva certezza sul buon esito degli articoli della Carta costituzionale, alcuni dei quali neppure a distanza di mezzo secolo hanno trovato concreta ed effettiva attuazione. ad esempio, all'articolo 39, che prevede la registrazione dei sindacati e il riscontro, elenchi degli iscritti alla mano, della loro consistenza numerica; ma potremmo rievocare grandi chimere come il proclamato diritto al lavoro o alla casa. L'accordo su un cambiamento di portata storica per il nostro Paese - e tale può definirsi la riforma di cui stiamo trattando - non può né trovarsi, né perdersi intorno ad aspetti che veniamo a definire strada facendo: un'intesa alta, come la richiedono le circostanze, nasce nel condividere la rotta di questo cambiamento. E quale sia la direzione a cui conduce il progetto di federalismo fiscale lo abbiamo indicato a più mani: si va, tra l'altro, verso l'autonomia impositiva degli enti locali; verso la compartecipazione ai tributi erariali e propri; verso la tracciabilità dei tributi, che consente al cittadino di giudicare del buon uso fatto dei propri soldi; verso il passaggio dalla spesa storica al costo standard per i servizi erogati; verso meccanismi di responsabilità per gli amministratori che maneggiano il denaro pubblico. Alla fine dei conti, per sovrammercato, ne risulterà la riduzione della pressione fiscale, auspicato effetto della modernizzazione nell'erogazione dei servizi e nell'ottimizzazione del rapporto costi-benefici, perché il sistema efficiente, tra gli altri, comporta il vantaggio di costare di meno. Colleghi senatori, enunciando tali misure provo la sensazione di elencare, in uno stretto rapporto di corrispondenza, principi come dignità, autonomia, sussidiarietà, correttezza, efficienza, onestà, parsimonia, senso di responsabilità e così via. Questi i valori del grande cambiamento che propugniamo; questa la piattaforma ideale intorno alla quale avremo potuto riconoscerci tutti con qualche entusiasmo di più. L'opposizione, invece, ha ritenuto di insistere sui nodi ancora da sciogliere, che pure vi sono, su criticità obiettivamente riscontrabili, ma da alcuni esposte in tono talmente perentorio da far ritenere che l'assenza di soluzioni preconfezionate e di pronta attuazione quasi possa minare l'intera impalcatura del provvedimento. È tuttavia in virtù dell'impegno da loro profuso in questa circostanza, e lealmente riconosciuto dal nostro movimento, che ci sentiamo di domandare ai colleghi del centrosinistra di fare comunque la cosa giusta, senza se e senza ma, guardando al significato prima che alla lettera della legge. D'altro canto, ci sentiamo di rassicurare l'opposizione sulle questioni sollevate: sollevate: il ministro Calderoli presenterà, in tempi brevissimi, una nuova e più organica versione della Carta delle autonomie, mentre il principio di perequazione viene recepito tra i cardini della nuova normativa. Quanto alla riduzione dei parlamentari, ricordo come questa scelta fosse già contemplata nella legge costituzionale che abbiamo visto passare senza esito al *referendum*. Dunque, chiediamo solo che si conceda tempo al tempo. tempo. Colleghi senatori, è durata vent'anni la lunga marcia della Lega Nord per portare a destinazione una riforma dello Stato in senso compiutamente federalista: la pazienza operosa e la sensata determinazione del nostro movimento dovrebbero parlare a chi ha orecchie e cuore per intendere. Parole a ragion veduta, perché non avremmo consentito che con un provvedimento raffazzonato, lacunoso o iniquo venisse sperperato il patrimonio di speranza e fiducia che la nostra gente ci affida e neppure che ne uscisse mortificata la diligenza dell'opposizione. Questo è l'impegno che la Lega Nord si assume davanti al Parlamento e al Paese.

Da esso, tuttavia, dobbiamo trarre anche elementi di ottimismo per il futuro, non senza rilevare alcune questioni che potrebbero mettere in crisi o indebolire questa fiducia

cattolica e quella liberale: il principio di sussidiarietà, avvicinare cioè il più possibile le istituzioni al cittadino ovvero cercare di valorizzare il più possibile l'attività dei cittadini, arretrando l'azione della mano pubblica. È un processo sofferto, certamente ben diverso da quello pensato dai Costituenti nel 1948: il regionalismo del 1948 indubbiamente una forma di decentramento molto attenuata e leggera rispetto a quella proposta nel 2001. A fronte di questi dati positivi, bisogna tuttavia svolgere alcune considerazioni il federalismo fiscale rappresenta l'altra faccia della medaglia del federalismo istituzionale, se non addirittura la stessa faccia in controluce.

abbiamo assistito a vicende di grande conflittualità e confusione. Fin dall'inizio, nel 2001, quando analizzammo la riforma introdotta in maniera affrettata dal centrosinistra, ebbi a rilevare che, di fronte a un federalismo pasticcione e confusionario, avrebbe vinto il più forte, e il più forte indubbiamente è lo Stato.

altrimenti rischiamo che anche il federalismo fiscale sia un federalismo di facciata, perché, a fronte delle contraddizioni e dei conflitti, vi sarà una vi sarà una fiscalità decentrata, rimessa ai livelli inferiori, ma non si realizzerà mai quella relazione tra potere, attribuzioni, competenze e responsabilità che un vero federalismo

è quella delle attribuzioni degli enti locali. La riforma degli enti locali non può più tardare perché, se arrivassimo ad attuare le norme delegate nel contesto attuale senza interventi razionali, logici ed efficienti sul piano delle attribuzioni, delle competenze e delle responsabilità,

dal complesso al semplice, dal decentrato all'accentrato, dal pluralismo tributario all'unicità del soggetto che imponeva i tributi, li gestiva, li regolava, li accertava e li esigeva (salvo alcune forme di decentramento sul territorio). Oggi questa riforma chiede di fare esattamente il contrario. E il contrario richiede, appunto, che vi siano soggetti titolari della potestà impositiva, della potestà accertativa e di quella di riscossione e che tali soggetti siano anche in grado di esercitare in maniera corretta le proprie funzioni per dare ai cittadini

tra potestà accertativa, potestà impositiva e ruolo e funzioni di carattere pubblico. I cittadini chiedono servizi, pagano le imposte

trasparente. Lo constatiamo di giorno in giorno, perché laddove si attribuiscono alle autonomie locali nuove potestà impositive, anche indirette, verifichiamo che i servizi non migliorano, ma aumenta il peso fiscale. Credo che ciò non sia nella volontà di chi di chi difende, sostiene e vuole portare avanti fino a risultati compiuti le norme contenute nel disegno di legge che ci accingiamo ad approvare in via definitiva in quest'Aula. *(Applausi

siamo autonomisti di vecchia data, con grande esperienza e abbiamo avuto la fortuna di poter vivere sul campo le vicende e i frutti di un'autonomia che significa nient'altro che una politica più vicina alla gente e più codecisa Pertanto, l'introduzione, o meglio (visto che è previsto dalla Costituzione) l'attuazione del federalismo fiscale, costituisce per noi una tappa per la modernizzazione del Paese, da realizzare tramite una formula importante:

costituenti hanno saputo gettare le fondamenta con un richiamo a principi liberali e democratici

non vale tanto per l'assetto organizzativo dello Stato. La struttura organizzativa e la divisione dei poteri da Stato centralista sono accompagnate da un timido regionalismo

Ci sono stati molti tentativi e li voglio ricordare in questa sede, perché stiamo facendo un passo in avanti in un percorso storico molto, molto sofferto. Le prime iniziative per dare a questo Paese un assetto più moderno e più vicino alla gente, più

grati a chi, poi, nonostante questi contraccolpi, ha promosso un passo in avanti.

per dare a questo Paese un assetto più moderno. Ricordo il vecchio filosofo Miglio, che già negli anni '90 aveva disegnato un'Italia con tre macroregioni, con il rispetto delle cinque Regioni speciali, per cui prevedeva uno statuto speciale. Ricordo però anche

testo della Costituzione ha modificato fortemente l'assetto del Paese: prevede il capovolgimento delle competenze residue a favore delle Regioni; prevede che la Repubblica non sia più "ripartita"

Pertanto, quello che stiamo approvando adesso è l'attuazione di una norma della Costituzione, dovuta e necessaria. Il disegno di legge prevede 24 mesi per la sua attuazione, responsabilizzando tutti i livelli di governo - amo ripeterlo - non solo per le spese, ma anche per le entrate, con l'auspicio di dare con ciò più responsabilità a tutto l'assetto finanziario del Paese,

Condividiamo quindi l'obiettivo di procedere alla graduazione e all'attuazione del nuovo quadro istituzionale: un passo in avanti verso uno Stato più moderno e più partecipato. Naturalmente, sappiamo tutti che i principi sui quali si basa il federalismo in Italia e anche in altri Paesi sono due. In primo luogo, l'articolo 119,

una perequazione sono in principio due, presenti in Europa e anche nell'economia politica: il primo è quello del federalismo cooperativo; il secondo è quello della competizione fiscale, che mette

i relativi strumenti come mezzo per migliorare la loro economia. Possiamo vedere questo strumento della competizione fiscale nella vicina Svizzera, dove i Cantoni lo

non raggiungeva neanche il 40 per cento della media nazionale. Nei trasferimenti dei fondi ha cercato poi di tener conto, per la metà,

infatti illuderci che soddisfacendo i princìpi base della Costituzione, cioè garantendo a tutti i cittadini uguali diritti

speranza che ciò porti a una riduzione e non a un aumento della spesa generale

Signora Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, oggi le tasse vanno a Roma e solo una piccola parte viene ridistribuita sul territorio. Con il federalismo fiscale, frutto della lunga battaglia di Umberto Bossi e della paziente azione diplomatica del ministro Roberto Calderoli, le risorse resteranno sul posto. Avremo un sistema premiante per Regioni ed enti locali che, a fronte di un alto livello dei servizi, offriranno una pressione fiscale inferiore alla media; previste al contrario sanzioni fino al commissariamento per chi sperpera i soldi pubblici. A trarre vantaggio dalla riforma sarà pure la lotta all'evasione fiscale: il coinvolgimento negli accertamenti degli enti locali, diventati beneficiari di una quota del prelievo, può rivelarsi un potente fattore di contrasto all'evasione. Inoltre, specie al Sud, troppo spesso i fondi pubblici, invece che generare sviluppo, sono finiti nelle tasche di qualcuno; ora i cittadini potranno controllare e, se è il caso, punire chi non amministra correttamente i loro soldi. Allo stato attuale nel nostro Paese su 100 euro di entrate tributarie ben 77,7 vanno all'Amministrazione centrale e solo 22,3 agli enti locali. In termini reali, a fronte di circa 459 miliardi di euro di entrate totali registrate nel 2007, all'Erario ne sono andati 357 e alle amministrazioni locali soltanto 102. Il centralismo fiscale italiano si traduce in una pressione tributaria di quasi 6 punti superiore alla federale Germania, il cui Governo centrale assorbe meno del 50 per cento di quanto versato dai contribuenti, e di 5 punti più alta della Spagna, che ha entrate centrali intorno al 55 Se si guarda poi alla competitività, l'Italia si colloca al 40° posto nel mondo, dietro a Paesi come Lettonia e Thailandia. A livello europeo siamo davanti solo alla Grecia. I dati emergono da un rapporto del centro di ricerca della rivista «The Economist»; secondo il periodico, la situazione italiana può però migliorare con il federalismo fiscale: una maggiore autonomia tributaria delle Regioni, se ispirata al principio della responsabilità, secondo cui il cittadino paga per ottenere un servizio, ne controlla l'erogazione ed esige la qualità dello stesso, renderà il servizio più efficiente. Il problema è nel modo di utilizzare le risorse: abbiamo quasi 60 dipendenti pubblici ogni mille abitanti, contro 55 di Germania e Spagna. Questo succede perché nella maggior parte dei casi chi lavora in istituzioni ed enti periferici è stipendiato dal centro. La pratica, frequente soprattutto nel Meridione, di assumere gli amici ha fatto lievitare oltre misura il numero dei dipendenti. Si tratta di un incremento che, dovendo pagare con i propri soldi, come avviene nei sistemi federali, non ci sarebbe stato. evidente che finché gli sprechi sono a carico di altri, anche se alla fine ci rimettono tutti, la situazione non cambia. In Germania, fra il 2000 e il 2007, la spesa per il personale pubblico, in percentuale del prodotto interno lordo, è scesa dall'8,1 al 6,9. In Italia, nello stesso periodo, i costi sono aumentati dal 10,4 al 10,7 per cento del PIL. Attualmente, quindi, siamo avanti di quasi 4 punti, con una spesa aggiuntiva di 60 miliardi di euro. Ad aggravare la situazione si aggiunge l'evasione fiscale. Uno studio dell'Agenzia delle entrate segnala nel nostro Paese realtà dove, ogni 100 euro dichiarati, ce ne sono addirittura altri 87 di reddito sommerso. Mancati introiti per lo Stato, che finiscono col tradursi in un ulteriore esborso a carico dei contribuenti onesti. Con l'autonomia fiscale gli enti locali avranno tutto l'interesse a recuperarli, creando un percorso virtuoso a vantaggio di tutti. «Se oggi», ha dichiarato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, «non si dà il senso di una forte capacità di autocritica e di autoriflessione nel Mezzogiorno, poi la partita per far passare politiche corrispondenti alle esigenze del Sud diventa enormemente difficile. Si possono denunciare rischi e paventare esiti infausti del federalismo fiscale, ma se ci si sottrae all'esercizio di responsabilità per quello che riguarda l'amministrazione della cosa pubblica nel Mezzogiorno, non si hanno titoli per resistere, anche alle interpretazioni più perverse del federalismo fiscale». Uno studio sul federalismo finanziario, fatto proprio dalla Conferenza dei Parlamenti delle Regioni d'Europa nell'ultima sessione di Bilbao, evidenzia come gli Stati federali abbiano costi di funzionamento inferiori (0,564 contro una media europea dell'1,000) rispetto a quelli centralisti. Il documento mette in mostra le grandi potenzialità dei modelli che prevedono sistemi fiscali e legislativi federali, dove in particolare la Svizzera rappresenta un esempio da seguire. Nella Confederazione elvetica ognuno dei 26 Cantoni, in qualità di Stato membro, gode di ampia autonomia, ha un proprio sistema scolastico ed un proprio Corpo di polizia. L'imposta federale è diretta e uguale per tutto il territorio nazionale, mentre l'imposta fiscale varia a seconda del Cantone e del comune, per cui vi è anche molta competitività poiché, com'è naturale, le persone e le imprese tendono a stabilirsi dove si pagano meno tasse. La Repubblica Federale di Germania è costituita da 16 *Länder*, simili alle nostre Regioni, che però hanno una propria costituzione, un'ampia sovranità e molti diritti di autonomia fra cui, pure qui, scuola e polizia. Il rapporto 2008 elaborato dalla Banca mondiale, che valuta la capacità dei singoli Paesi di favorire o inibire l'attività imprenditoriale misurando l'apparato amministrativo, organizzativo, fiscale, legale, economico e finanziario, conferma l'efficacia dei sistemi federali, collocando la Svizzera al sedicesimo posto su 178 Paesi, il Belgio al diciannovesimo, la Germania al ventesimo, l'Austria al venticinquesimo. L'Italia è cinquantatreesima, seguita in Europa solo da Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia e Grecia. *(Applausi

signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'esame di questo disegno di legge in materia di federalismo fiscale l'Italia dei Valori apprezza il fatto che per la prima volta, dall'inizio della legislatura, sia stato seguito un *iter* legislativo che ha consentito di analizzare nel merito il contenuto del provvedimento e le proposte emendative presentate. è stato un paziente lavoro, una cultura dell'ascolto che, purtroppo, nella prassi di questo primo anno di legislatura che festeggiamo domani, è mancata tra maggioranza e opposizione. Ci auguriamo che l'impianto del disegno di legge sul federalismo fiscale possa portare ad una cultura della responsabilità

È stato già ricordato che abbiamo un debito pubblico elevatissimo, 1.700 miliardi di euro, che nonostante l'abbattimento dei tassi di interesse è destinato ad aumentare e non a diminuire; un debito che grava per 28.000 euro - cito a memoria - su ognuno dei 60 milioni di abitanti: qualcosa come 78.000-80.000 euro per ognuno dei nuclei familiari, e l'impianto di questa legge deve portare alla riduzione delle spese e non certamente ad un loro aumento. Cito brevemente alcuni articoli che sono stati anche il frutto degli emendamenti e della cultura del dialogo, dell'ascolto e anche del lavoro svolto dal Gruppo Italia dei Valori nelle Commissioni riunite e in Aula, sia alla Camera dei deputati

(o il fabbisogno) standard sia assunto quale costo (o fabbisogno) che dovrà valorizzare l'efficienza e l'efficacia al fine di costituire l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica. Vanno, inoltre, definiti gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni indicate nella norma. 2, dell'articolo 2 richiede che i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici siano individuati in modo da assicurare la redazione dei bilanci di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in base a criteri predefiniti ed uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata, coerenti con quelli che disciplinano la redazione dei bilanci. L'articolo 2, comma 2, lettera *i)*, prevede l'obbligo di pubblicazione - anche questa è un'innovazione - sui siti Internet dei bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, tale da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite* secondo modelli uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata. Voglio ricordare che proprio oggi la procura della Repubblica di Milano ha emesso un'ordinanza per sequestrare a quattro banche banche circa 465 milioni di euro. Queste banche estere (Deutsche Bank ed altre) avevano appioppato strumenti derivati.

non vi sia da parte degli enti locali, magari poco responsabili, la possibilità di addossare alle future generazioni, per 30 o 40 anni, i debiti

sottolineo quell'emendamento, presentato nel corso dell'esame in sede referente, che dispone che ciascuno schema sia corredato da una relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico. La lettera *c)* dell'articolo 7, riformulato nelle Commissioni riunite, ha specificato che per una parte dei tributi propri previsti da leggi statali le Regioni possono variare le aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale e nel rispetto di quella comunitaria. Le Regioni possono altresì modificare con propria legge le percentuali delle aliquote delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla normativa statale. L'articolo 26 reca i criteri per la definizione di un sistema premiale e sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultano virtuosi o meno rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti. Il sistema sanzionatorio che si applica nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica comporta molti divieti. Le sanzioni indicate si applicano fin tanto che l'ente non metta in atto i provvedimenti necessari in grado di riportare l'ente medesimo in linea con gli obiettivi di finanza pubblica. L'articolo 28,

di copertura finanziaria degli oneri relativi alla costituzione e al funzionamento degli organi di cui agli articoli 4 o 5, ossia rispettivamente la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Infine, l'articolo 28, comma 4, reca la clausola di copertura finanziaria ai sensi della quale dal provvedimento in esame e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il contenuto degli ultimi due commi dell'articolo 28 recepisce l'emendamento dell'Italia dei Valori presentato in sede referente alla Camera dei deputati.

resti fermo il principio ai sensi del quale il Governo, in allegato al primo schema di decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore legge - dovrà trasmettere alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Chiudo, signor Presidente, onorevoli colleghi, augurandomi che questi emendamenti possano trovare accoglimento e auspicando che, a un anno dalla legislatura, la cultura del dialogo e dell'ascolto, la pazienza del ministro Calderoli e la pazienza anche nostra nelle Commissioni possano essere replicate nel prosieguo della legislatura. Di fronte a una crisi sistemica come questa, infatti, lo scontro per lo scontro e, magari, anche proposte di riforma

alla storia per convincersi di come prodursi nell'azione politica attinente il futuro, si potrebbero nutrire forti perplessità sulla giustezza di quello che stiamo facendo, non tanto perché esiste

per l'altra notazione che viene dalla conoscenza del passato, e cioè che la ricchezza dei precedenti ci può confortare nell'azione relativa al futuro. per l'unità d'Italia, di cui anche quest'Aula è piena di richiami con le iscrizioni bronzee alle spalle di codesta Presidenza,

Cosa invece ci può confortare che così non è? Il fatto che tutti abbiamo imparato che si governa meglio se il programma delle parti politiche procede secondo i desideri dei propri elettori, provvede alle necessità del popolo governato e ricerca il consenso per quello che si dice e si fa non soltanto dei propri elettori, ma di quanti più elettori possibili e, quindi, anche di chi ha votato la parte competitrice. Allora, ci potrebbe lasciare pensare il fatto che, in definitiva, questo provvedimento non riceve grandi critiche neanche da parte dell'opposizione in ordine ai contenuti sostanziali. Ci sono riserve rispetto alla Carta delle autonomie e rispetto alla possibilità che questo provvedimento abbia un costo e che nessuno dica quanto potrebbe

quando questa parte politica, rispetto alla parte competitrice ancor più alfiere del provvedimento, si dice convinta del provvedimento stesso, lo fa

soltanto agli elettori della Lega in Lombardia e in Veneto, ma anche a tutti gli altri di Forza Italia e di Alleanza Nazionale. Cito la Lombardia perché, sin

come la Lombardia, che hanno un residuo attivo molto elevato. Se gran parte della popolazione si ritiene nelle condizioni di versare all'Erario molto di più di quello che riceve, è chiaro che quella parte della popolazione ritiene anche che una trasformazione in senso

che tenta di equilibrare le discrasie che provengono dal prelievo fiscale e dalla utilizzazione dello stesso.

una contrapposizione di programmi e di princìpi, cioè una contrapposizione politica, se si tiene conto che questo sistema può essere la salvezza del Mezzogiorno.

che nel momento in cui esiste una Comunità europea fortissima, a questo punto gli Stati hanno perso di significato. Queste stesse persone potrebbero essere anche quelle che abitano nel triangolo industriale

Ci salva il fatto che, se ci cimentiamo in una trasformazione della forma di Stato, per cui è lo Stato centrale a mediare rispetto agli egoismi territoriali,

subito dopo il famoso *referendum* confermativo della riforma costituzionale approvato il 7 ottobre 2001 dal popolo italiano. Mancano i numeri

casa. Il federalismo che ho in mente è fatto di autonomia e responsabilità, due parole che non si possono scindere. È troppo semplice spendere i soldi che arrivano dall'alto. Molto più difficile è spendere i soldi che l'amministratore locale deve chiedere ai cittadini.

Signora Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, nel 2011 ricorreranno i 150 anni dall'Unità d'Italia; è una storia giovane di una Nazione che inizia ad esistere 200 anni fa con Napoleone. Paradossalmente, l'unico tentativo di un embrione di storia nazionale fu avviato, neppure consapevolmente, da un popolo germanico che invece proprio certa storiografia nazionalista risorgimentale additò al pubblico disprezzo: i Longobardi. Finito il *regnum* *Langobardorum* alla Chiusa di San Michele, terminò anche la possibilità di dare all'Italia un'autentica tradizione nazionale. È noto, infatti, che di Nazione italiana non si può parlare per l'esperienza romana: i cittadini di *Mediolanum*, *Perusia*, *Neapolis*, *Brundusium* erano cittadini romani di originaria *natio* celtica, etrusca, greca, illirica; erano del resto romani, almeno a partire da una certa epoca, al pari di quelli di *Lugdunum* (Lione) o di *Vindobona* (Vienna). Cosa caratterizza dunque la nostra storia? Noi siamo un insieme di popoli di culture e origini diverse ma con una unità di valori, una civiltà che si ispira ad un comune filo conduttore, che è poi quello romano e cristiano; aggiungerei un'unità di sensibilità. L'Italia è una sorta di Stati Uniti *ante litteram*, cioè il Paese che ha fatto *ex pluribus, unum*. Vi sono alcuni periodi gloriosi nel nostro passato: certamente, quello romano. L'esperienza romana fu caratterizzata da un eccezionale strumento di autogoverno: il municipio. La romanizzazione della penisola italica passa attraverso i municipi che avevano proprie leggi, una propria giurisdizione, una propria amministrazione, originariamente persino una propria moneta. I territori italici, che non erano annessi e organizzati nelle forme del municipio, erano uniti a Roma da *foedera*, patti, che rappresentavano la forma originaria del moderno federalismo. L'altro grande periodo fulgido della nostra storia è certamente quello dei liberi Comuni. E poi l'Umanesimo e il Rinascimento, dove peraltro le repubbliche e le signorie erano veri e propri stati sovrani con ciascuno una propria politica estera. La nostra è dunque una storia plurale, fatta di straordinarie ricchezze, una storia non banalmente, grigiamente omogenea, ed eguale, ma una storia di differenze. La nostra è una unità nella diversità. Dunque l'idea federale è quella che più si adatta alla identità del nostro Paese, l'unica che consente di costruire una Nazione che non sia un'immagine caricaturale o un Moloch opprimente ma una realtà viva e feconda. Il federalismo fiscale che ci apprestiamo a varare è solo un aspetto, importante ma strumentale. È cioè uno strumento di qualcosa che deve essere più ampio e, comunque, è solo un punto di partenza. Di certo non è, per esempio, il modello svizzero o quello tedesco. Nel modello svizzero i Comuni e i Cantoni sono autosufficienti. Non è il modello spagnolo,

Auspicabilmente, si potrà incidere sul cosiddetto residuo fiscale, quel famoso residuo fiscale che ha creato molto malumore e molte sperequazioni nel nostro Paese. introduce per la prima volta nel nostro sistema il principio di responsabilità: anche questo è un passo avanti importante. L'obiettivo vero, però, è quello di arrivare ad un modello di federalismo istituzionale che vada oltre la riforma del 2001 e che superi, peraltro, le impostazioni della stessa *devolution*, che operava entro una operava entro una cornice indifferenziata e che per questo, soprattutto al Sud, fu rifiutata. Il vero federalismo di cui ha bisogno il nostro Paese è differenziato, secondo uno *slogan* che si potrebbe riassumere come "a ciascuno secondo le sue necessità". È questo il modello seguito in un altro Paese che ha una storia plurale alle spalle, come la Spagna. È il modello degli Statuti di autonomia particolare. Dirò subito che per certe Regioni italiane una forte autonomia è, allo stato attuale, persino pericolosa e negativa. In certe aree del Paese ci vuole più Stato. Ovviamente, deve essere uno Stato che faccia solo quello che serve, uno Stato autorevole e non inquinato da camorre e mafie di vario genere. Altre Regioni potrebbero invece già ora gestire in proprio una serie importante di competenze ulteriori. Faccio degli esempi concreti: la scuola, innanzitutto. Regioni come la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Toscana e altre ancora possono senz'altro gestire in proprio non solo l'istruzione professionale, ma anche l'istruzione tecnica e l'istruzione tecnica superiore. Ciò significa che per questi settori anche la formazione, il reclutamento, l'organizzazione scolastica, i programmi, lo stato giuridico dei docenti dei settori specifici che ho nominato possono passare a quelle Regioni che siano in grado di gestirli efficacemente. può essere oggetto di devoluzione a quelle stesse Regioni il diritto amministrativo dell'impresa, vale a dire il regime delle autorizzazioni e delle concessioni, ma anche l'organizzazione sanitaria, alcune regole nel settore del mercato del lavoro, la bassa giurisdizione in campo civile ed in specie l'organizzazione dei giudici di pace, la tutela del decoro degli ambienti urbani fino alla previsione di norme di natura penale, l'organizzazione giuridica del territorio. Occorre altresì introdurre albi regionali degli insegnanti che, pur conservando il carattere nazionale dell'abilitazione all'insegnamento, impediscano i consueti fenomeni di transumanza interregionale, che lasciano scoperti perennemente gli organici di certe Regioni. La crisi del contratto nazionale è evidente. I sindacati devono capire che ciò che conta non può essere l'interesse delle nomenklature di confederazione. Ai lavoratori non interessa il destino di quanti segretari generali perderebbero peso e ruolo da una progressiva localizzazione della contrattazione. Ai lavoratori interessa che il potere d'acquisto dei propri salari sia meglio garantito. È assurdo che un tranviere o un insegnante non possano declinare le proprie condizioni contrattuali tenendo conto delle specificità economico-sociali locali. Il sindacato non ha ancora risolto il problema della territorializzazione della rappresentanza e della contrattazione. Infine, occorre un Senato delle Regioni che ponga termine al bicameralismo perfetto,

non si può non istituire una Corte con una composizione che tenga conto delle Regioni, magari attingendo a quel terzo che oggi è espresso dalle magistrature. Non esiste Paese al mondo in cui la Corte costituzionale sia espressione della magistratura (peraltro di correnti della magistratura), cioè non soggetta al principio della sovranità popolare. No al governo dei giudici, sì al governo del popolo, popolo che va inteso anche nelle sue articolazioni territoriali. Questa Repubblica dovrà essere cementata da un Presidente eletto da tutti gli italiani,

cui contenuti fondamentali, quali la partecipazione, il coinvolgimento dal basso - come è nello spirito della Lega - di tante istituzioni, enti ed organismi, sono la testimonianza vera e tangibile di quanto odierna, attuale, moderna e sempre attenta al territorio sia l'attività politica della Lega.

essere capaci di scegliere il meglio di ciò che gli altri possono proporre, ovvero le famose *best practices* di cui tanto si parla anche in tante attività industriali.

una coincidenza tra centro di spesa, di responsabilità e di entrata, in modo tale che non vi sia quella confusione che regna adesso all'interno delle nostre istituzioni, per cui non si sa più chi fa che cosa e a chi ne risponde.

anticipando quella che è una grande necessità di riordino e di trasparenza, nella logica della pulizia di tante leggi inutili che da subito, come sta facendo bene

fare delle riflessioni che vanno nel senso di dare delle risposte ad una serie di osservazioni che soprattutto l'opposizione muove rispetto a questo provvedimento. È certo che ci siamo intrattenuti sulla definitiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, perché nel 2001 si è voluto riformare la Costituzione nel modo improprio che tutti quanti noi sappiamo. E quelle critiche che oggi vengono mosse dalla sinistra sulla mancata attuazione degli articoli 114, 117 e 118 vanno nel segno di un impianto riformatore e innovativo realizzato a colpi di maggioranza, ma che non rispondeva ad un organico disegno di riforma complessiva della Costituzione. Si è voluti intervenire, ad esempio, sulle competenze del sistema delle autonomie, delle Regioni e degli enti locali, senza bilanciare i poteri dello Stato e senza pensare alla forma di Governo. Sicché tutte le obiezioni che vengono mosse riguardano poi il merito di alcune competenze, che sono state al centro di motivazioni ostative di contrapposizione che la sinistra ha mosso negli anni precedenti al nostro disegno di riforma costituzionale. Riguardavano, ad esempio, la competenza sulla pubblica istruzione o sulla polizia sulla polizia locale e, più estesamente, alcune competenze che in questi anni, nella contrapposizione con la competenza concorrente hanno determinato di fatto un blocco delle attività complessive in svariati ed importanti

Oggi puntiamo a realizzare quanto è scritto nella Costituzione attraverso una possibile legge di delega, e riteniamo che ci siano una serie di risposte da dare che non possono essere risolte unicamente, così come si richiede, trovando analogo momento di applicazione per quanto stabilito negli articoli 114, 117 o, meglio ancora, 118 si sta lavorando con il Testo unico degli enti locali e la riforma complessiva di quel settore strategico e nevralgico, in particolare per quanto riguarda alcune competenze. Ma c'è un problema più generale che riguarda

quella che impropriamente viene definita una applicazione del federalismo fiscale, ma che è una riforma che interesserà principalmente il sistema delle autonomie (e attendiamo l'altro pezzo, su cui stiamo lavorando:

tutta quella nuova classe dirigente, soprattutto degli enti locali, che si va formando nel Mezzogiorno d'Italia e che in questi anni ha dovuto sopportare il ruolo preponderante delle Regioni come centro di spesa e non come centro di legislazione secondaria. Vi è anche la grande questione del centralismo regionale che opprime il sistema delle autonomie locali, che non trasferisce risorse, che è incapace di progettare, di delegare verso il basso le competenze e che assegna agli enti locali un ruolo marginale, soprattutto perché non dispongono di risorse adeguate. A tal proposito,

Ma una riflessione è necessaria. Questo impianto, che verte sulla responsabilità diretta di chi sul territorio deve amministrare le pubbliche istituzioni, deve essere collegato agli altri contrappesi che dobbiamo predisporre, esempio la necessaria riforma del sistema delle autonomie, tenendo presente che non bisogna partire dalla criminalizzazione della politica. Molto spesso ci lasciamo

a lei, in particolare, l'impegno, l'attenzione, la disponibilità al confronto e alla modifica del testo legislativo che ha dimostrato per tutto l'*iter* parlamentare di questo progetto di legge al Senato, alla Camera e poi di nuovo al Senato.

invece che questa disponibilità venga mantenuta in tutto il percorso di approvazione dei decreti attuativi, in cui sarà decisivo il lavoro della Commissione bicamerale. Lei ben sa, signor Ministro, che è nei decreti attuativi la sostanza vera del federalismo che intendiamo realizzare nel nostro Paese.

inopportuno normare il federalismo fiscale, dando attuazione all'articolo 119 della Costituzione, senza avere ridefinito l'assetto delle competenze e delle funzioni delle autonomie locali; senza aver riscritto, in sostanza, la Carta delle autonomie locali.

della norma sull'abolizione dell'ICI sulla prima casa ha determinato un credito da parte dei Comuni nei confronti dello Stato di oltre un miliardo di euro, ma determina anche grandissime difficoltà nella finanza comunale. I tagli realizzati in settori strategici, quali la scuola, la sanità, l'assistenza, l'edilizia scolastica (che ricadono in modo molto significativo sulla vita delle famiglie e sugli enti locali), sono gravissimi proprio per le loro ricadute sulle comunità locali. Ricordo inoltre le elargizioni del tutto arbitrarie in favore del Comune di Catania, 140 milioni di euro, e nel Comune di Roma, pari a 500 milioni di euro, e la scelta di non aver voluto allentare i vincoli del Patto di stabilità neppure per i Comuni "virtuosi", che hanno disponibilità finanziarie molto significative e che potrebbero investirle con estrema rapidità per migliorare i servizi destinati alla loro comunità e per dare impulso allo sviluppo economico e all'occupazione. C'è dunque grande incoerenza tra

Io penso esattamente il contrario: sono proprio questi i momenti che richiedono una grande coesione da un lato, ma anche una grande capacità di riforma. Oppure, signor Ministro, si tratta di una politica condivisa e studiata: la politica delle enunciazioni di principio a cui non seguono fatti coerenti.

Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il tema del federalismo fiscale ci ha occupato a lungo

e anche di colloquio e di dialogo tra parti, che forse su altri temi non riescono ad intendersi e che invece su questo hanno trovato il modo di comprendersi. svolgere un intervento un po' problematico, dato che alcuni colleghi toccheranno, con maggiore precisione, gli aspetti più tecnici. Vorrei anzitutto mettere in rilievo una sorta di problematicità del contesto in cui si vengono a trovare il provvedimento in esame ed il nostro stesso modo di affrontarlo. C'è un aspetto di natura pubblicitaria che non va trascurato e che in qualche modo è anche giustificato. Questo provvedimento infatti è sostanzialmente intestato alla Lega

Noi lo abbiamo inteso soprattutto come occasione da gestire con sapienza per riuscire a determinare un maggiore controllo delle comunità sui volumi di spesa. quella che è stata chiamata anche da altri colleghi la prassi della responsabilità, l'evidenza fondamentale del principio di responsabilità: accede a questo ragionamento sulla spesa non più come una massa di cittadini intesi come clienti che si aspettano i vantaggi dati dallo Stato; si invece, ad una prassi per cui le comunità e i territori si interrogano sulle effettive risorse a loro disposizione esercitando una presa di coscienza.

l'esperienza del passato non è straordinariamente ottimistica, cioè non ci induce molto all'ottimismo. Ricordo, di passaggio, che la faticosa attuazione delle Regioni ha costituito - tra tante altre cose che possono essere considerate positive e significative - una gigantesca espansione della gigantesca espansione della spesa ed anche una moltiplicazione delle strutture amministrative burocratiche; il decentramento del governo nel territorio ha prodotto enti

consulenze, appalti e l'enorme rigonfiamento del materiale amministrativo. Insomma, le Regioni rappresentavano l'attuazione di un principio costituzionale e, quindi, bisognava farle. però, una rilettura autocritica del modo con cui le Regioni si sono costituite potrebbe salvarci anche dal rischio di ricadere nello stesso errore.

Certamente le Regioni hanno costituito un formidabile impulso all'aumento dei costi della politica e bisogna evitare che la prassi del federalismo fiscale aggiunga qualcosa in questo solco.

una logica che postula o postulerebbe - secondo alcuni più, secondo altri meno - la necessità di aggiustamenti nell'architettura istituzionale: istituzionale: la collega Bastico ricordava giustamente la necessità di mettere a punto una Carta delle autonomie, che ancora non c'è; si deve fare un ragionamento sulla modifica del bicameralismo perfetto. In proposito, si apre un orizzonte che non è detto si debba guardare con fervente ottimismo. Ho davanti uno schema mentale che sento ripetere moltissimo dappertutto, dagli organi di stampa, dal Governo e da molti protagonisti della scena politica, per cui, di fatto, il federalismo fiscale chiama come conseguenza istantanea il complesso ridisegno del bicameralismo perfetto, la trasformazione del Senato in una qualche cosa che è, comunque, una Camera delle Regioni.

di questa ipotetica unità nazionale frazionata sotto lo sguardo benevolente di un Presidente eletto direttamente, con tutto quello che comporta in termini di modifica costituzionale. Considero questo tipo di prospettiva nefasta. Penso che sarebbe infinitamente più saggio ragionare in termini di realizzazione,

questo tipo di processo produca un frazionamento dell'unità nazionale e considero del tutto fuori dal mondo la possibilità che si possa ricomporre l'unità nazionale nella maniera retorica della riconduzione del tutto ad un Presidente unificante. Quello che succede nella prassi politica ha depositato già qualche tossina su questo piano:

come se dovesse essere sostituito da un rapporto plebiscitario tra capo e popolo. Ci sono segni, anche nella prassi quotidiana, di questo processo e li considero assolutamente negativi.

quando viene a parlare della necessità di riforme dice che è incombente l'argomento del rafforzamento dei poteri del *Premier*.

il *premier* Berlusconi ha un potere speciale e aggiunge che quando Berlusconi uscirà di scena, se non saranno intervenute modifiche costituzionali, torneremo rapidamente alla regola italiana dei Capi di Governo deboli. Francamente, vista la forza, preferisco un Capo del Governo debole rispetto all'esibizione di una forza scomposta. Ma il punto fondamentale che viene a giorno è il seguente: se già abbiamo di fronte un *premier* più più forte di quello che dovrebbe essere, non si vede perché dovremmo immaginare un'architettura istituzionale che, presumibilmente, a questo *premier* si appresta a consegnare un sovrappiù di potere, ulteriormente rafforzato e sostenuto,

Penso che sarebbe molto saggio se ragionassimo in termini progressivi e costruttivi sulla costruzione effettiva del federalismo fiscale, lasciando veramente da parte questa sorte di proiezione inquietante che getta una luce distorcente su tutti i processi di modifica istituzionale. Il collega Valditara si è spinto persino a dire che dentro questo quadro di unificazione plebiscitaria perfino la Corte costituzionale dovrebbe subire una torsione e non mi sembra un buon segno che si incomincino ad elencare addirittura le conseguenze secondarie del rafforzamento di un potere dell'Esecutivo ultradimensionato. Abbiamo lavorato insieme discutendo di federalismo fiscale ed il giudizio, nel complesso, suffragato anche dall'accoglimento di alcuni

Il giudizio positivo non è un giudizio positivo preventivo. Saremo attentissimi a valutare il modo con cui i decreti attuativi trasformeranno in prassi le scelte di sistema.

la lealtà istituzionale tra i diversi livelli di governo, la necessità della trasparenza dei bilanci, la progressività dell'imposizione fiscale, che in Italia praticamente non esiste, il controllo delle Camere sul rapporto tra Governo e pareri parlamentari. C'è, invece, una grande opacità sulla questione della logica dei rapporti tra Regioni e Comuni, evidenziata anche da altri

Province e Città metropolitane diventano una nuova occasione di moltiplicazione, dispersione e dissipazione di risorse pubbliche. C'è il passaggio dalla spesa storica al costo standard e l'esigenza però di

*(PdL)*. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il federalismo di cui parliamo oggi, e su cui domani voteremo per la seconda volta, facendo sì che esso diventi finalmente legge della Repubblica, non è quello di Carlo Cattaneo, né quello di Luigi Einaudi; non ha alle spalle una violenta guerra mondiale, né dolorose scelte fratricide. Il federalismo di cui parliamo oggi non ha un proprio Manifesto di Ventotene, ha alle spalle intellettuali come Altiero Spinelli, Ernesto Rossi o, per legarlo al concetto di autonomia tanto caro ai colleghi del Movimento per l'Autonomia, come Mario Alberto Rollier, il quale pensava ad un federalismo che partisse dalle autonomie regionali, forse per esorcizzare il pericoloso ritorno di pericolosi nazionalismi. Il federalismo di cui parliamo oggi non passa per le grandi, ma lente e complesse, svolte costituzionali, che pur devono essere compiute, ma attraverso il desiderio impetuoso di un Paese stanco di subire la sua stessa inefficienza, stanco dei suoi ritardi e dei tradimenti compiuti e subiti. Il nostro è un Paese che ha voglia di coniugare, in maniera armonica, termini come sussidiarietà, efficienza, solidarietà, equità, ma anche responsabilità, trasparenza, senso dello Stato, economia di scala. Per lanciare il Paese verso questa nuova epoca, verso questa nuova dimensione, dopo quello che sono stati il fascismo, il comunismo, la guerra, il dopoguerra, il piano Marshall, la Cassa per il Mezzogiorno e - perché no certi errori di Garibaldi e Bixio e dell'intera dinastia savoiarda, la storia ha scelto questo Parlamento, questo Governo e il suo *leader* Silvio Berlusconi. Come alla fine di un ballo mascherato, cominciato a metà dell'Ottocento, oggi con questa legge vengono tolte le maschere: si può guardare bene il volto dei danzatori e capire chi è stato vittima e chi carnefice, chi ha costruito l'Italia e chi l'ha distrutta, chi ha usato lo Stato per acquisire consenso e chi, invece, lo ha servito.

sin dalla loro costituzione, possa rappresentare un modo attraverso il quale bloccare il sistema e soprattutto eludere la perequazione infrastrutturale. Ha ragione, il rischio c'è, ma non la sua fondatezza, dato che dietro l'azione di un Esecutivo che volesse fare il qualsiasi colore esso sia, c'è sempre un Parlamento ed un elettorato pronti ad intervenire smascherandolo. Il federalismo fiscale non è un traguardo, è una tappa. Non può esserci federalismo fiscale che non produca un federalismo politico ed un federalismo partitico, come accade nella Catalogna o nei Paesi Baschi e come non può che accadere anche nel nostro Paese. Non può esserci federalismo fiscale senza perequazione infrastrutturale e senza che, per tempo, vengano saldati i conti sociali, strutturali, territoriali, soprattutto quelli vecchi. Nel corso del mio intervento, svolto in occasione del primo voto su questa legge, accennai a quello che hanno rappresentato per il Sud 150 anni di politiche unitarie ed oltre 60 anni di democrazia repubblicana.

delle patate, il 41,5 per cento dei legumi, il 60 per cento dell'olio. Nel 1861 la razione di carboidrati per abitante del Sud era di 418 grammi, contro i 270 grammi delle altre parti del Paese. Pensate che il 55 per cento della forza lavoro in agricoltura ed il 51 per cento della forza lavoro nell'industria era al Sud, e non c'era la cassa integrazione, così come erano al Sud i due terzi delle riserve auree del Paese. La prima ferrovia, la prima illuminazione a gas, il primo corpo dei vigili del fuoco furono realizzati al Sud. Il Sud, a quel tempo, ha sfamato il Nord impoverendosi, come è accaduto anche con i provvedimenti anticrisi che ribaltano le emergenze. Il Sud ha permesso alle corti, prima monarchiche e poi repubblicane, di sprecare le sue risorse all'interno di un quadro centralistico devastante, ma adesso il ballo mascherato è finito e i conti su chi deve dare e chi deve avere o li farà il Governo - e li farà certamente - o temo che li faranno i cittadini. Quei cittadini del Sud, ma anche del Nord, spesso tenuti in letargo da una classe politica inetta, parassita o ascara a cui quei conti dovranno essere mostrati con tanto di certificazione contabile e di efficacia. E in quei conti (rispondo al collega Stradiotto e sottolineo che ha ragione il collega Ferrara), dovranno esserci sia le pensioni di invalidità, sia le ore di cassa integrazione, sia i chilometri di autostrade, sia il numero di aule scolastiche, sia i chilometri di ferrovia, sia il numero e la qualità degli ospedali, sia le arance dell'AIMA, sia le quote latte, sia i dipendenti pubblici delle Regioni rosse, sia le promozioni di massa fatte in Sicilia dai Governi a guida PDS alla fine degli anni Il federalismo fiscale è una tappa alla quale i ministri Calderoli e Bossi hanno molto lavorato sotto la vigile guida del Presidente del Consiglio, ma anche il Parlamento ha fatto la sua parte e deve continuare a farla con attenzione e rigore

troppi Comuni e troppi consiglieri inutili, troppe Province in cerca di competenze, troppi enti mangiasoldi nati per collocare clienti e funzionari di partito, troppi ATO spreconi e inefficienti, troppi istituti autonomi case popolari che gestiscono senza risolvere. In questo Paese ci sono troppi consigli di quartiere senza deleghe, troppe cariche duplicate, troppi parlamentari, troppi organismi che governano i medesimi territori, sovrapponendosi, complicando la vita dei cittadini e sprecando le risorse dello Stato. Il federalismo fiscale deve significare smascherare gli strumenti di una falsa democrazia sprecona e acquisitiva, ma anche gettare via l'acqua sporca contenuta in questi organismi, salvando e ridistribuendo le loro competenze, se non sono solo solo figlie della burocrazia e del burocratismo. Se lo sono, invece, buttando via anche quelle. So che il Governo sta lavorando in questa direzione e, dunque, sono fiducioso che presto un'altra tappa nel percorso di modernizzazione dello Stato verrà compiuta. Mi rendo conto che non sarà facile, ma so che è necessario. Per vedere gli effetti, come consiglia Schopenhauer, dobbiamo fare come con un mosaico: "Da vicino non se ne colgono i particolari, le immagini non suscitano impressione, è da lontano che bisogna guardare per trovarle belle e significative". non dobbiamo pensare, come cinici politicanti, alle prossime elezioni, compiendo scelte funzionali a coltivare clientele e bisogni che spesso passano attraverso le ignobili vie della democrazia acquisitiva, dobbiamo pensare ed operare da statisti su cui pesa la responsabilità non solo dell'oggi ma anche del domani. Ecco perché federalismo fiscale deve significare anche demolizione di un sistema democratico fondato troppo spesso sulla gestione delle necessità dei deboli e dei bisognosi e costruzione di un nuovo sistema democratico fondato sulla trasparenza, sull'efficienza, sulla competenza, sul merito, sulla passione e sull'onestà. Mi piacerebbe parlare dell'impatto non fiscale, né economico di questa legge, bensì dell'impatto sociologico e politologico ma il tempo è tiranno e non bisogna approfittare della generosità di quei poche che ascoltano. Dunque, concludo auspicando che il percorso politico ed istituzionale intrapreso in questi mesi continui, illuminato non da una lanterna ma dal sole, così che esso possa rivelarci ogni dettaglio, ogni necessità, ogni strada e non solo la solita strada. A chi ha contestato la via ordinaria e non costituzionale verso il federalismo e a chi, in mancanza di altri argomenti, l'ha giudicata inadeguata o, addirittura, immorale, sfoggiando tutto il pessimismo di cui è portatore, potremmo rispondere con due citazioni. La prima è di don Lorenzo Milani, il quale diceva che «al mondo i valori più grandi si raggiungono col minimo di mezzi». La seconda è di Filippo Turati, il quale sosteneva che «la ferocia dei moralisti è superata soltanto dalla loro profonda stupidità». È per questo che noi andiamo avanti, fiduciosi nell'intelligenza dei cittadini e nella loro enorme capacità di capire, sempre e bene, ciò che gli accade intorno e di decidere per il meglio.